Rispetto a circostanze precedenti, nelle quali la 5a Commissione si era riunita per assolvere allo stesso compito, abbiamo preso atto del fatto che il Governo non ha apportato alcuna modifica modifica rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati ed esaminato dalla Commissione nel corso della discussione generale sul provvedimento. La riunione della Commissione ieri sera è stata, quindi, la sede per la riproposizione, da parte della maggioranza e da parte dell'opposizione, degli argomenti già affrontati nel corso della discussione generale e già richiamati, signor Presidente, nel mio intervento ieri mattina in Aula, nel quale ho dato conto

essere riferita al disegno di legge di assestamento, così come invece può avvenire per gli oneri determinati dal provvedimento per il 2007. In sostanza, colleghi, l'opposizione

sia scorretta, ma il tasso di lontananza rispetto all'applicazione corretta della legge di contabilità si accresce - secondo l'opposizione - quando ci si riferisce alla copertura degli oneri determinatisi con il decreto per gli anni 2008 e 2009.

per la previsione di copertura degli oneri 2008 e 2009 il riferimento non può essere all'assestamento, ma deve essere necessariamente ai quadri tendenziali di finanza pubblica

sto sempre riferendo della tesi dell'opposizione - non è una norma e non può in nessun caso essere preso a base per recare mezzi di copertura per una legge che comporta oneri ulteriori. Fin qui la tesi dell'opposizione, che spero di aver riferito correttamente. Posso soltanto aggiungere, signor Presidente, che in ogni caso e qui invece riferisco della mia opinione e non di quella dell'opposizione - per la prossima legge finanziaria bisognerà avere grandissima cura nel controllare - dovrà farlo il Governo soprattutto, ma certo il ruolo del Parlamento su questo punto dovrà essere decisivo - che il miglioramento del risparmio pubblico per il 2008 e il 2009, tassativamente, possa essere utilizzato a copertura, facendo riferimento al suo importo netto, cioè al suo importo una volta sottratti i mezzi di copertura copertura sul 2008 e sul 2009, che vengono utilizzati da questo decreto per coprire gli oneri riferiti a quegli anni. Infatti,

La maggioranza, invece, per parte sua, ha insistito - come già ho avuto modo di riferire ieri su argomenti di fatto - li chiamerei così - riferendosi, per la copertura degli oneri recati dal decreto,

questo è l'argomento che risponde alla tesi precedente dell'opposizione sui mezzi di copertura riferiti al 2008 e al 2009 - al carattere strutturale degli incrementi di entrate, tali cioè da riproporsi anche negli anni successivi. Quindi, quello della maggioranza è stato, mi si consenta, un argomento in via di buona sostanza, e cioè: è vero è vero che vi sono problemi sotto il profilo della forma, ma le entrate stanno aumentando davvero; in una quota rilevante questo aumento di gettito è di tipo strutturale, per cui non stiamo facendo correre, in buona sostanza, alla finanza pubblica alcun rischio particolare perché siamo in un ambito di assoluta tranquillità sotto il profilo del carattere strutturale degli aumenti di gettito che si stanno determinando. Lo stesso andamento delle entrate 2007 - questa, in sostanza, è la tesi della maggioranza - conferma che siamo in presenza di un aumento strutturale, così da fornire anche per il 2008 e il 2009 ampie garanzie sull'effettiva copertura degli oneri determinati dal decreto-legge, peraltro minori, per quegli anni, rispetto a quelli che si determinano per opera dello stesso decreto-legge per il 2007. In ogni caso - questo è l'ultimo argomento - l'assestamento 2007 e il bilancio di previsione 2008 forniranno, anche sotto il profilo formale, quella copertura che oggi viene garantita in via di sostanza. Questo è stato, grosso modo, l'andamento della discussione in Commissione sui profili di copertura finanziaria del decreto-legge. Spero di aver riportato, con una certa puntualità e correttezza, le tesi opposte,

riferendomi ai precedenti, intervenire. Il presidente Morando ha svolto la sua relazione ed è uso - perché non è regolamentato - che l'opposizione, in ordine a quanto riferito, dica qualcosa. In questo senso non so se dovermi riferire al Regolamento o all'ordine del lavori,

per segnalare semplicemente all'Aula che si sta consumando, grazie a quanto illustrato dal presidente della

ho il piacere d'intervenire all'inizio di questa seduta dopo la breve, ma significativa, relazione del presidente della al quale però vorrei ricordare che definire strutturali le maggiori entrate e dare per certo e per scontato che anche negli anni futuri si realizzeranno,

Solo la settimana scorsa la maggioranza di questo Senato ha approvato un DPEF dal respiro brevissimo, molto attento agli interessi politici immediati e poco attento agli interessi di finanza pubblica e, in generale, del Paese. È stato definito dai più autorevoli commentatori economici, spesso persino dell'area culturale e politica di questa contraddittoria maggioranza, un DPEF di fine legislatura, sostanzialmente elettorale. È un po' come se voi sapeste di dover tornare presto al giudizio degli elettori e, come è vostro costume, cercate di raccogliere consenso allargando a dismisura i cordoni della borsa. E lo fate con risorse che non avete nemmeno contribuito a creare, poiché con le vostre politiche non si creano risorse, le si consumano. Quel famoso "tesoretto" che vi siete ritrovati tra le mani grazie ad una fase positiva dell'economia della zona euro e soprattutto all'azione lungimirante del Governo Berlusconi in materia fiscale e di rientro dal *deficit,* non è vostro, è degli italiani. Voi, invece che sfruttare il ciclo positivo, preferite prendere tempo (o meglio perdere tempo) su tutto: riforme strutturali, pensioni, mercato del lavoro, riforma fiscale, contenimento della spesa pubblica. Il DPEF ha rinunciato a realizzare ciò che poteva essere fatto e probabilmente ha ragione Giulio Tremonti quando chiarisce che gli italiani sono il vero "tesoretto" del Governo Prodi dei senatori a vita. Infatti, sono sempre loro a pagare, pagare, pagare... Non serviva molto, bastava ascoltare i consigli del Fondo monetario, dell'Unione Europea o meglio ancora della Banca d'Italia e della Corte dei conti, che suggerivano una semplice strategia economica che qualsiasi cittadino di buon senso applica alla propria famiglia, nella propria impresa:

si cambia la giacca, chiude nel cassetto le analisi e fa il Ministro della spesa. Il Ministro ha, infatti, fatto tutto il contrario di ciò che asseriva a Bruxelles: ha deciso di spendere quei 6,5 miliardi di euro, invece dei 2,5 più volte annunciati, e dimenticato nel cassetto, quello dove aveva riposto le analisi, ogni aggiustamento al bilancio del 2008. Va capito il Ministro: tiene famiglia, e anche grande. Tra comunisti, ex comunisti, neocomunisti, comunisti confessionali, similcomunisti e comunisti verdi non deve essere facile. Hanno vinto un gratta e vinci, questo è il

Scusate il paragone un po' semplicistico, ma, secondo me, rende bene l'idea della vostra politica economica, tesoretto più, tesoretto meno. Ciò significa che l'aggiustamento previsto per la finanziaria 2008 sarà pari a zero, mentre il *deficit* per il 2008 sarà rivisto al rialzo al 2,2 per cento. Per la prima volta, dopo tanti anni, gli obiettivi sono peggiori del tendenziale. La strada quindi verso il raggiungimento del pareggio di bilancio è comodamente rinviata al 2009, al 2010, al 2011, fosse per voi, all'eternità. Con buona pace di comunisti, ex comunisti, neocomunisti, similcomunisti, comunisti confessionali e comunisti verdi. Un pessimo segnale quello che avete dato in questi giorni di banchetto a Palazzo Chigi. Il Ministro del Il Ministro del Governo Prodi dei senatori a vita aveva promesso riforme vere e non selvaggi tagli di spesa, ma tra DPEF e decreto fiscale non si vedono né le riforme, né i tagli, ma solo la vecchia logica della spesa pubblica sospinta dalle tasse, e quando le entrate aumentano la spesa pubblica finisce sempre per aumentare. Per le riforme poi c'è sempre tempo. tempo. Dopo, quindi mai. Di sicure ci sono solo le spese, tante spese. Complimenti al ministro Ferrero, che ha strappato quasi 2,5 miliardi di euro per interventi aggiuntivi in campo sociale. Peccato che non lo faccia con soldi virtuosi, frutto di eliminazione di sprechi, ma sempre con lo stesso trucchetto: più tasse più spese, più spese più tasse, dov'è la carta è qui la carta. Ve lo hanno dimostrato le analisi del senatore Baldassarri e dell'economista Renato Brunetta, persino quelle di Nicola Rossi indicano che i vostri conti sono truccati. Ha ragione Brunetta: gli atti parlamentari su questo tesoretto dovrebbero essere trasmessi e costituire formale denuncia del Governo Prodi dei senatori a vita alla Corte dei conti. Ecco perché Prodi ha invocato "l'ingerenza" della Chiesa, che dalle sue omelie domenicali aiuti questo strampalato Governo a ficcare bene nella testa degli italiani che devono pagare di più, ogni anno di più. E al vice ministro Visco, che è venuto in Commissione bilancio a spiegarci la natura di questo extragettito, definendolo, leggo dal resoconto per essere precisa "dovuto

ascrivibile non alla riduzione della pressione fiscale", avvenuta negli anni passati durante il Governo Berlusconi "ma ad un crollo degli adempimenti spontanei dei contribuenti in previsione dei condoni attuati dal Governo precedente", quel Governo Berlusconi che non ha mai legiferato considerando i propri cittadini sudditi e utili solo a pagare le tasse. Veda, vice ministro Visco, ella può anche non venire in Parlamento

in controtendenza con il resto dell'Europa e con il resto del mondo. Il ministro Padoa‑Schioppa spieghi agli italiani che forse è più bravo a fare le analisi economiche, piuttosto che aiutare questa nostra economia traumatizzata da continui elettroshock di *deficit spending* dell'allegra compagnia di comunisti, ex comunisti, neocomunisti, similcomunisti, comunisti confessionali e comunisti verdi.

l'ennesimo salasso agli italiani, agli onesti lavoratori italiani, ai giovani italiani, alle donne italiane, alle famiglie italiane, alle imprese italiane. Grazie, senatori a vita, scivolerete con *nonchalance* tra i velluti del Senato e, un po' sordi per scelta e un pochino per l'età, non riuscirete ad udire il lamento del popolo italiano, che anche di voi non ne può più.

all'Aula e alla Presidenza, sull'articolo 1 di conversione del decreto all'esame dell'Aula, hanno un significato non regolamentato, come nell'altro ramo del Parlamento, ma introdotto per decisione della Presidenza nel corso della precedente legislatura.

ai sensi di cosa intervenire, se del Regolamento o dell'ordine dei lavori. La motivazione dell'intervento è quella di ripetere, ancorché la comunicazione del Presidente della Commissione bilancio sia stata stata resa nel miglior modo possibile (e di questo lo ringraziamo), e sottolineare un elemento in più che non può essere contenuto nella relazione del Presidente. Il Presidente della

a conforto non soltanto del contenuto del testo, ma anche a conforto dell'ammissibilità dell'articolo. A nostro avviso, quindi, resta comunque

la responsabilità dell'ammissibilità. A questo punto volevamo sottolineare e far rimanere a verbale che a nostro avviso la Presidenza sta ammettendo un decreto giuridicamente scoperto. Perché questa aggettivazione? Come ha spiegato il presidente Morando, è stata fatta una distinzione tra la sostanzialità e la

che è formalmente scoperto, ma, poiché la formalità nella contabilità avvolge la sostanzialità, questo significa che è anche sostanzialmente scoperto.

se in futuro non si terrà conto del già utilizzato miglioramento del risparmio pubblico, si utilizzerà due volte tale risparmio e quindi - *mutatis mutandis* - è come se si stesse gestendo in dirittura di fallimento lo Stato. È questo il motivo per cui ci

una legge di contabilità, quindi con l'ordinamento giuridico che deve contenere l'autorizzazione delle risorse dello Stato, di fatto, non ci consente di determinare la sostanzialità della copertura, in quanto, ripeto, (e a questo punto bisognerebbe riferirsi a concetti filosofici, ma che si possono benissimo trasporre in politica e in matematica finanziaria) il contenuto ha significato soltanto se vi è una forma che l'avvolge.

tre riflessioni, e spero di essere breve, su questo provvedimento che davvero è stato, per gli italiani, un tormentone. Oggi finalmente il tormentone finisce, questo *refrain* del tesoretto ci lascia. Non ci lascia però questa maggioranza che del tesoretto ha fatto una questione francamente imbarazzante. Circa un anno fa, di questi tempi, si era di fronte ad uno scenario che gridava al dissesto fino al rischio di uscire dall'Europa a causa di un debito stratosferico. Oggi siamo invece così ricchi da non sapere come spendere il tesoretto. Al Governo che si è impegnato in un dibattito estenuante e lacerante sulla consistenza di questa manovra

dal Governatore della Banca d'Italia e da tante altre autorità e organismi che provvedono al controllo del sistema economico, che hanno raccomandato al Governo di utilizzare tali risorse per il risanamento dei conti pubblici, con scelte politiche rigorose, mediante un approccio strutturale. Il Governo, invece, si è distinto per perseguire obiettivi di spesa polverizzati, quasi degli *spot* di spesa, piccoli interventi riconducibili ai consumi intermedi.

da una tassazione per qualche verso vessatoria cui i cittadini del nostro Paese sono sottoposti. Egli rilevava, inoltre, un incremento della pressione fiscale dal 40,6 al 42,3 per cento, insostenibile e incompatibile con politiche di sviluppo, certo unica possibilità per politiche di spesa diffusa e disarticolata che non hanno alcuna valenza strategica, come quelle che questo Governo ha scelto e determinato. Ho ascoltato la collega Bonfrisco e mi pare sia giudizio diffuso l'incertezza sulla strutturalità di queste entrate e quindi la necessità di un loro utilizzo razionale, non estemporaneo, che potesse in qualche modo contenere esigenze diverse. Forse era opportuno che il tesoretto segnasse la conclusione della stagione della finanza creativa e quindi, per esempio, servisse a recuperare quella operazione dissennata quale il dirottamento del TFR all'INPS, misura che sta scoraggiando il decollo della previdenza integrativa ed è un buco contabile che maschera l'andamento effettivo dei conti pubblici, la vera lezione da trarre dal miracolo del 2006 è che la mancata trasparenza è un'arma a doppio taglio. Tra l'altro, il miglioramento dei conti è derivato non da un contenimento della spesa, e questo provvedimento ne acuisce le caratteristiche di largheggiamento, ma, appunto, da maggiori entrate. Vorrei provocare il Governo, perché non ho una cultura rigorista in economia e non sono appassionato alla rigidità dei vincoli di bilancio. Forse per una giovanile formazione keynesiana immagino che un intervento pubblico, una mano pubblica che sovrintenda alle scelte macroeconomiche sia legittima per affrontare nodi e vincoli strutturali di un Paese. Quindi, è perfettamente legittimo se un Governo ha la forza di assumere l'iniziativa di rendere maggiormente flessibile la manovra di bilancio, di rinviare nel tempo, con uno scadenzario meno rigoroso, il rientro dal debito, con scelte che facciano respirare di più la comunità, attraverso stimoli significativi al sistema economico. Ma il fallimento di questo provvedimento è proprio nel non avere accettato questa sfida, nel non aver utilizzato le risorse dell'extragettito per un'operazione legittima anche dal punto di vista della politica del consenso: quella di rilanciare il sistema economico attraverso interventi mirati sui nodi che aggrediscono lo sviluppo del Paese, sulle infrastrutture,

di innescare processi virtuosi di crescita strutturale del nostro sistema economico. Perdonatemi, vi sembrerà una tiritera ed un *refrain* anche il mio, visto che ne parlo continuamente, ma ognuno di noi assolve ad una funzione in un ambito parlamentare. Gli elettori della mia circoscrizione mi hanno affidato il compito di ricordare e di sollecitare costantemente il tema mancato dello sviluppo del Mezzogiorno. Quanto

e delle infrastrutture da allocare nell'area meridionale. Le sofferenze e le povertà, di cui tanti amici e colleghi della sinistra antagonista si menano, ricordando in questa sede un valore insopportabile per il nostro Paese, sono allocate lì, in quelle aree: è lì che risiedono le sacche di povertà e di emarginazione; è lì che

della disinvoltura, della disattenzione che questa compagine di Governo rivolge a quell'area territoriale e politica. c'è anche il valore di una classe dirigente politica che si misura nella capacità di imporre i temi dello sviluppo di un'area. Tale tema tema dovrebbe attraversare trasversalmente questo emiciclo e l'altro della Camera, e forse anche la compagine di Governo, per produrre iniziative *bipartisan* che assumano

del CNEL. Non c'è un solo soggetto, in nessun ambito scientifico e culturale, che studi questa area territoriale che non colga le drammatiche condizioni di emergenza sociale. Però, il Governo questo non lo ha fatto. Il Governo, come ha detto ieri un collega, piuttosto che governare il Paese, si preoccupa di governare la sua maggioranza; si preoccupa di governare i dissidi, le tensioni nobilmente, diremmo - la dialettica di una maggioranza composita e frammentata. La vicenda del tesoretto è il paradigma di questa condizione e ne costituisce alla fine il postulato anche la questione di fiducia. Ieri ho ascoltato il ministro Chiti motivare le ragioni che hanno indotto il Governo a porre la questione di fiducia. Non vi era, proprio per il carattere estenuante di questa

è un elemento inaccettabile, per due ragioni. Anzitutto, se la maggioranza fosse davvero compatta non si sottrarrebbe alla sfida parlamentare. luogo, definire intangibile un provvedimento del Governo che viene presentato al Parlamento è un'offesa alle prerogative parlamentari e alla normale dialettica Governo-opposizione. La verità, e concludo, è che il profilo della sfida tra le componenti - e la questione delle pensioni appare come fonte di grande inquietudine per il Governo il Governo - li ha consigliati di rinviare la partita a settembre e di chiudere frettolosamente e ignominiosamente questa stagione di Governo, segnata dall'inconcludenza e dall'incapacità.

maggioranza in un solo anno di Governo. Per cui, nei prossimi mesi di vita che restano alla maggioranza e al Governo, probabilmente si riuscirà a superare anche questo record e a porre

di lavoro amministrativo ha, di fatto, perso sostanzialmente la fiducia di tutti gli italiani, soprattutto di quella parte che magari aveva creduto in questa maggioranza e nel suo programma e l'aveva votato un anno fa. E il Governo ha perso la fiducia non in maniera casuale ma proprio per gli interventi che ha adottato in quest'anno. Quindi, prima di parlare di questioni economiche, in particolare della

al mondo della magistratura e soprattutto introduceva princìpi che in realtà dovrebbero essere cardini ideologici di questa maggioranza, almeno a sentire le cose che dice, introducendo un minimo di meritocrazia, un minimo di avanzamento di carriera in base all'effettivo impegno del giudice, un minimo di chiarezza nella

in quel decreto, dal momento che poi, alla fine, il grande risultato economico per il Paese è stata la fantomatica liberalizzazione dei tassisti, con conseguente abbattimento delle tariffe (tant'è che prima del decreto

nella finanziaria 2007, al punto che ormai, come abbiamo visto tutti in questi mesi, la maggior parte delle aziende non lavora più per avere un minimo di utili da reinvestire,

aumentando drasticamente la contribuzione per gli apprendisti. In tutto è arrivata una settantina di nuove iniziative fiscali con conseguenti appesantimenti

l'evasione fiscale, presente in alcune aree del Paese dove tutta la filiera industriale è in nero, obbligando le aziende che già sono regolari, pagano le tasse ed hanno tutti i libri contabili in regola, ad aggiungere il

o si sono spesi 30 miliardi in più di spesa corrente o c'è qualcos'altro che non quadra. Ricordo semplicemente che l'extragettito è il risultato fiscale dell'anno precedente, mentre la spesa è il risultato economico della gestione dell'anno scorso. In realtà, quindi, si tratta di ha sperperato 30 miliardi di extragettito in un anno e che non ha saputo indicare nessuna strada alternativa per lo sviluppo economico del Paese; un Paese che cresce la metà del resto d'Europa

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto‑legge sul maggior gettito tributario, così com'è impostato dal Governo, rappresenta un'autentica delusione per tutti i cittadini italiani ma, segnatamente, per quelle fasce sociali più deboli del Mezzogiorno, dei lavoratori dipendenti, delle famiglie e delle imprese. Si tenta di ridurre la pressione fiscale utilizzando maggiori entrate senza che queste siano state mai iscritte al bilancio. È prevista una spesa ulteriore di 7 miliardi di euro senza avere le relative entrate. C'è il rischio reale, in autunno, di predisporre una nuova manovra aggiuntiva di almeno 15 miliardi di spesa. Com'è ben evidente, la crisi economica sarà ancora più marcata e la competitività del nostro apparato produttivo sarà sempre più flebile rispetto ai nostri diretti competitori europei. Il Commissario europeo per gli affari economici ha, infatti, espresso profonda preoccupazione per la scelta del Governo italiano e del ministro dell'economia Tommaso Padoa-Schioppa di realizzare per il 2008 e per gli anni successivi un consolidamento inferiore a quanto promesso a Bruxelles. una decisione che il Commissario ha definito «non in ottemperanza con gli orientamenti dell'Eurogruppo del 20 aprile» scorso, in cui si chiedeva di corregge il rapporto *deficit*-PIL dello 0,5 per cento annuo e di destinare tutto l'extragettito al risanamento del Paese. La sinistra di Governo non ha ancora spiegato come ridurre il *deficit*, né come ridurre il debito, né come migliorare la qualità della finanza pubblica con simili provvedimenti che sono velleitari, inconcludenti e demagogici. Il decreto Bersani, unica e sola vera perla di questo Governo, è veramente punitivo, quasi una vendetta sociale nei confronti dei ceti medi produttivi, dei commercianti, degli artigiani, dei tassisti, dei farmacisti, dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi. Noi riteniamo che le proposte avanzate sulla destinazione del tesoretto non vanno a colmare né a risarcire i sacrifici dal popolo italiano sino ad oggi. Siamo in presenza di un Governo irresponsabile che lascia nel vago molte importanti riforme, rinviando tutto alla legge finanziaria per evitare così ulteriori lacerazioni nella maggioranza governativa prima delle vacanze estive. In autunno, però, il presidente Prodi saprà che tutti i problemi non affrontati porteranno sicuramente alla crisi politica, una crisi di una maggioranza divisa su tutto; non c'è strategia economica; ci sono forti divaricazioni di ordine sociale; ci sono forti penalizzazioni e forti ritardi nelle infrastrutture per le aree più deboli del Paese. Voglio solo ricordare che il Governo Berlusconi aveva approvato la legge obiettivo e ripartito con una programmazione rigorosa le grandi opere infrastrutturali in tutte le aree del Paese; il Governo Prodi, invece, di fatto ha cancellato quella programmazione ed ha rimesso in circolazione una serie di interventi a pioggia finalizzati solo ad accontentare questa o quella forza politica, questo o quel senatore per mantenere unita questa traballante maggioranza. Per esempio, signor Presidente, da calabrese prima e da parlamentare dopo, mi piacerebbe mi piacerebbe avere delle serie motivazioni sulla fine che hanno fatto i 450 milioni di euro destinati alle infrastrutture viarie della Calabria. Assieme a venti colleghi senatori della Repubblica ho presentato un'interpellanza urgente ai Ministri competenti per capire che fine avevano fatto i soldi che il Governo Berlusconi aveva stanziato per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Fino ad oggi nessuna risposta è pervenuta da un Governo incapace, persino, di mantenere rapporti corretti con il Parlamento della Repubblica. Devo ricordare che nella legge finanziaria 2007 è previsto, all'articolo 1, uno stanziamento di 150 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 per un totale di 450 milioni di euro da utilizzare per gli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità di competenza delle cinque Province calabresi. La norma prevedeva che con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con quello dello sviluppo economico, si provvedesse alla ripartizione di tali risorse tra le Province della Regione Calabria. Nel corso di alcuni incontri il ministro Di Pietro illustrava i contenuti della norma prima richiamata e richiedeva alle amministrazioni provinciali uno sforzo per la definizione dei programmi di investimento e della conseguente progettazione esecutiva. Il ministro Di Pietro in un ulteriore incontro tenutosi in Calabria, in provincia di Cosenza, garantiva ai sindaci di quella Provincia il fondo per l'attuazione di infrastrutture viarie per la finanziaria 2006. A questo incontro, egregio Presidente, seguirono dichiarazioni roboanti e trionfalistiche da parte del Presidente della Giunta di sinistra della Calabria e del Ministro competente, il quale affermava che i fondi sarebbero stati disponibili entro il 30 giugno 2007. Successivamente, però, agli stessi rappresentanti regionali convocati a Roma è stato comunicato dal Ministro che «dei 450 milioni destinati alla Calabria non c'era traccia nei capitoli della Finanziaria». Siamo, come è del tutto evidente, in presenza di un'azione a dir poco truffaldina, fatta sulla pelle di una Regione che ha già di per sé gravi problemi di ordine sociale ed economico. Signor Presidente, si accertino le responsabilità e mi auguro che ci siano anche delle conseguenti decisioni politiche per coloro i quali si sono resi responsabili di simili misfatti. In ogni caso questo decreto, cosiddetto tesoretto, così come il DPEF, non prevede nel capitolo infrastrutture alcuna somma da poter utilizzare per rilanciare l'economia del Mezzogiorno: nessun cenno alle somme abusivamente sottratte a questa parte del Paese! Anzi, il capo del Governo Prodi, insieme ai verdi ed ai rifondaroli di casa nostra, ha affermato ripetutamente in Calabria che i fondi accantonati da Fintecna per la costruzione del ponte sullo Stretto andavano utilizzati per definire opere primarie in Calabria. Sino ad oggi siamo in presenza, ancora una volta purtroppo, di atteggiamenti politici irresponsabili che al danno aggiungono la beffa: non avremo il ponte sullo Stretto, non avremo potenziate nemmeno le strade della Calabria. Vorrei ricordare, infine, che questo Governo è stato eletto soprattutto per i voti determinanti dei calabresi, dei lucani, dei pugliesi, dei campani. Ma queste popolazioni, sino ad oggi, dal Governo Prodi hanno ricevuto solo mance, solo profonde delusioni che hanno accresciuto le distanze siderali che già esistevano tra elettori ed eletti. Nessun cenno è stato fatto alle emergenze meridionali: il 25 per cento delle famiglie vive sotto la soglia di povertà; nel Sud d'Italia il 50 per cento dei giovani è disoccupato, 500.000 famiglie monoreddito sono alle prese con l'emergenza abitativa degli affitti, per cento degli edifici scolastici non è a norma di legge per quanto attiene la sicurezza. Il Mezzogiorno d'Italia insomma è fortemente deluso ed amareggiato e ha buon diritto di protestare e richiedere un nuovo voto politico, con nuove elezioni, che tendano a spedire definitivamente a casa un Governo insipiente, incapace, sordo a tutte le aspettative delle popolazioni amministrative meridionali.

Signor Presidente, mi consenta di esordire con una nota di carattere personale; purtroppo non c'è il ministro Chiti, al quale avrei chiesto se poteva cortesemente scusarsi con me per aver ieri storpiato il mio nome nel rispondere alle osservazioni che ho fatto in sede di dibattito generale. Signor Presidente, il problema può sembrare di poco momento, perché in fondo - per così dire - sono anche consapevole di avere un cognome complicato che talvolta può essere difficile da pronunciare in prima battuta. Però è come cittadino italiano e non come senatore (questo è fatto accidentale della mia vita e non sostanziale) che mi sono sentito in qualche modo non rispettato a sufficienza dal mio Governo, perché il diritto al nome e all'identità della persona in fondo è qualcosa di importante ed è anche rivelatore, in chi si preoccupa di chiamare gli interlocutori con il loro nome, un segno che distingue lo stile e la creanza

alla discussione sulla fiducia. Ebbene, se in questo Paese esistesse la possibilità, per l'opposizione, di adire la Corte costituzionale per la legittimità costituzionale degli atti del Governo, le cose che ha detto ieri il ministro Chiti a giustificazione della questione di fiducia Ieri contestavo un fatto preciso a cui il Ministro non ha risposto, forse perché nella concitazione del poco tempo che avevamo a disposizione non mi sono riuscito a spiegare con sufficiente chiarezza. Come dicevo, se esistesse la possibilità di adire la Corte, le parole del ministro Chiti - che adesso vedo in Aula seduto tra i banchi della maggioranza e quindi penso mi possa anche ascoltare - sarebbero state - sarebbero state il cuore di una memoria dell'opposizione per chiedere la decadenza dell'atto formale che lui ha posto in essere. Infatti, ieri il Ministro ci ha detto che la fiducia è stata posta non perché esistesse un ostruzionismo dell'opposizione, che certo non poteva manifestarsi essendo stata posta la fiducia molto tempestivamente non esistessero ragioni di altra natura che lo giustificassero, di verifica interna alla maggioranza), ma semplicemente per fare in fretta, perché il Governo vuole che questi provvedimenti entrino in vigore il prima possibile. Ebbene, mi permetto di rilevare che la nostra Costituzione assegna una potestà legislativa di carattere assolutamente eccezionale e straordinaria al Governo e precisa in due articoli, nel 76 e nel 77, come si esercita tale facoltà assolutamente straordinaria ed eccezionale, ponendo dei limiti invalicabili per quanto concerne la possibilità del Governo di sostituirsi al Parlamento nel legiferare con la decretazione di urgenza.

entri in attuazione in tempi utili. Utili a cosa? Utili a far crescere, a far tornare un po' in alto il consenso perduto da questo Governo? Utili a che cosa? Non c'è una ragione costituzionale

che ha fatto della difesa della Costituzione del '48 una trincea invalicabile e ha mobilitato il Paese in un una occasione referendaria costituzionale affinché la Costituzione del '48 fosse salvata (mi chiedo dove sia quel sepolcro imbiancato del presidente Scalfaro, con i suoi farisaici appelli a salvare la Costituzione) ci passeggi ora allegramente sopra per ragioni meramente elettoralistiche e di convenienza politica. È qualcosa che dovrebbe provocare indignazione in coloro i quali sono sostenitori strenui della difesa della Costituzione e dei suoi valori. Ma si sa, la doppia morale è la morale e la doppiezza è l'essenza dell'essere e questo è il motivo unico per il quale si può porre la fiducia in quest'Aula con argomenti che costituzionalmente provocano orrore e disgusto. Chiunque abbia un minimo di decenza istituzionale e costituzionale dovrebbe reagire

come noi, ha cercato di cambiare, secondo le legittime procedure, la Costituzione di questo Paese e ha continuato ad accusarci di essere eversori costituzionali, accetta come normalità che si ponga la fiducia su questo provvedimento per le ragioni che il Ministro ha detto ieri in quest'Aula. Se esistesse un minimo di dignità e di sussulto costituzionale in quest'Aula, tutti i colleghi ieri avrebbero dovuto reagire, per dire che non è questo il modo in cui si tratta il Parlamento, non è questo il modo in cui si tratta il Senato. Devo ringraziare, a questo proposito, il presidente della Commissione bilancio, senatore Morando, per l'onestà intellettuale con la quale ieri, nell'illustrazione

Sono oltremodo ulteriormente indignato per il fatto che il Ministro non abbia sentito neanche l'esigenza di rispondere ai puntuali rilievi che il Presidente della Commissione, che incidentalmente è anche membro della sua stessa parte politica, ha svolto in quest'Aula richiamando tutti noi ai doveri e alle prerogative del Parlamento e del Governo. Detto questo - e già basterebbe per bocciare la fiducia al Governo, che fa della Costituzione quel che gli pare e che gli viene comodo all'uso, salvo poi ammantarsi di essere il difensore delle istituzioni e dello spirito repubblicano - è incredibile la commedia degli equivoci e delle ipocrisie

il punto non è che il Governo abbia posto la fiducia a sorpresa, ma il contrario: la fiducia era annunciata da tempo, era stata posta anche alla Camera, quindi si sapeva perfettamente che questo sarebbe accaduto. Il punto è, signor Presidente, che si è atteso per porre la fiducia formalmente il momento preliminare alla fase della discussione e del voto sugli emendamenti. Onestà intellettuale avrebbe voluto che il Governo la ponesse subito, all'inizio della procedura. Se abbiamo un problema di credibilità delle istituzioni rispetto ai cittadini e le polemiche di questi mesi sulla casta di cui faremmo parte ‑ e a cui non mi sento francamente di appartenere

sin dall'inizio il coraggio di dire «il Parlamento non discuta neanche un minuto, il provvedimento è prendere o lasciare», forse avremmo avuto maggiore chiarezza e non avremmo avuto titoli come quelli sui giornali di oggi:

Sul merito, come ho già detto ieri, questo è un provvedimento che denota tutta la cultura politica e di politica economica della sinistra, la quale ha massacrato gli italiani raccontando regalie. Il Presidente del Consiglio, dopo aver mentito due volte sullo stato dei conti pubblici aver assunto l'impegno a non aumentare le tasse e averlo smentito alla prima legge finanziaria, oggi pensa di salvarsi la coscienza con qualche regalia, facendo ingoiare anche ai colleghi di Rifondazione il rifinanziamento delle missioni all'estero a cui sono contrari.

*(Aut)*. Signor Presidente, questo provvedimento rappresenta una prima risposta alla nostra mozione approvata in quest'Aula con la quale abbiamo chiesto al Governo un cambiamento di rotta nella politica fiscale. È un provvedimento che va nella direzione giusta; è il primo provvedimento che corregge l'indirizzo di politica fiscale al quale devono necessariamente seguirne altri. Il Paese ne ha bisogno. Il provvedimento contiene *in* *toto* misure a favore dei cittadini tali da riuscire finalmente a dare un segnale di alleggerimento del peso fiscale e prevedere interventi di tipo socio-economico molto attesi da una vasta platea di contribuenti. Mi riferisco, in particolare, all'aumento delle pensioni minime dei soggetti più disagiati, o alle norme sulle percentuali di deducibilità delle spese per le auto aziendali e ad altre disposizioni che correggono misure previste dalla legge finanziaria per il 2007 come, ad esempio, gli alleggerimenti burocratici a favore delle piccole imprese e del volontariato. Inquesto senso vanno la disposizione che esonera i soggetti in regime di contabilità semplificata e le associazioni di volontariato dall'obbligo di presentare l'elenco clienti-fornitori per l'anno 2006 e la disposizione sugli indici di normalità economica, disposizioni che sono state inserite dal Governo nel testo del decreto- legge e che riprendono due nostri emendamenti concordati qui in Senato con maggioranza e Governo durante la trattazione del disegno di legge n. 1485.

una precisazione molto importante al fine di eliminare ogni equivoco interpretativo e dare certezza di diritto ai contribuenti. La norma contenuta nell'articolo 15, comma 3-*bis*, elaborata anche in accordo con le categorie, estende agli indicatori di normalità economica il carattere di presunzione semplice, la non automaticità degli accertamenti e l'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria già in vigore per gli studi di settore, così come previsto dall'articolo 62-*sexies* 30 agosto 1993, n. 331, e dall'articolo 2727 del codice civile e inoltre confermato dalla giurisprudenza. Durante la trattazione di questo argomento alla Camera sono state espresse, da alcuni colleghi, perplessità nel senso che la formulazione della norma sugli studi di settore potrebbe essere interpretata a sfavore dei contribuenti. È proprio per ovviare a queste preoccupazioni e per garantire la corretta applicazione della norma che in Commissione finanze abbiamo espresso un parere favorevole al provvedimento, a condizione che sia chiarito (è proprio questo il chiarimento che sto chiedendo adesso) che sia per gli studi di settore che per gli indici di normalità economica valgono la presunzione semplice, la non automaticità degli accertamenti e l'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria. In tal senso ho anche presentato l'ordine del giorno G15.100 (testo 2), che purtroppo non potrà essere votato perché è stata chiesta la fiducia. Mi aspetto quindi che il Governo in replica faccia la precisazione richiesta nel senso appena auspicato, proprio per garantire la certezza del diritto e l'applicazione corretta della volontà del legislatore. colleghi, questo provvedimento rappresenta una svolta nella politica fiscale attuata fino ad ora e ringrazio il Governo per aver accolto le sollecitazioni da noi fatte in quest'Aula. Non ci possiamo permettere errori nella politica fiscale. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio che ci permetta da una parte di combattere efficacemente l'evasione fiscale e dall'altra di contenere la pressione fiscale e gli obblighi burocratici. Dobbiamo seguire Dobbiamo seguire la politica fiscale adottata dai Paesi europei a noi più vicini iniziando a ridurre la pressione fiscale e a semplificare gli adempimenti amministrativi perché dobbiamo reggere la concorrenza internazionale. I contribuenti vogliono un fisco più equo, un fisco che combatta l'evasione fiscale, ma che non si ostini a colpire solo determinate categorie o in modo più insistente certe aree geografiche. Siamo tutti consapevoli del fatto che l'evasione è fortemente presente nel Paese: combattiamola con imparzialità e controlli mirati che siano equamente distribuiti sul territorio nazionale: è la migliore tutela del contribuente onesto.

contenuto nell'articolo 53 della Costituzione, in base al quale "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". il principio di un rapporto di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione finanziaria nell'osservanza delle norme contenute nello Statuto del contribuente.

inversione di tendenza nell'attività del Governo; anzi, notiamo con sempre maggiore preoccupazione i salti che sta facendo rispetto alla linea del famoso rigore che aveva annunciato e da cui in ogni momento si discosta, per cui non riusciamo più a capire la filosofia del bilancio e della manovra finanziaria di questo Governo. Ci viene chiesta la fiducia: ma come facciamo a dare la fiducia ad un Governo

dati statistici recentissimi dicono che nei prossimi due anni, se non cambia qualcosa, 1.700 imprese sono a rischio, anzi, chiuderanno sicuramente.

di fronte ad una risorsa straordinaria, per la quale per fortuna non dobbiamo chiedere sacrifici a nessuno in quanto già esistente, e non la si utilizza per dare risposte alle difficoltà effettive che conosciamo. conosciamo. Si abbandona la politica di rigore. Abbiamo due Ministri che montano ogni giorno sul piede di guerra, salvo poi lanciare non più *ultimatum* ma *penultimatum,* perché sembra che l'*ultimatum* vero non ci sia assolutamente. Il Governo continua a giocare: un giorno si risana e il giorno dopo si ridilapida. A noi sembrava che, condivisibile l'iniziale posizione del Governo, dovendo rientrare dal debito,

Prendiamo atto che probabilmente questa manovrina, che si spalma su alcuni soggetti, può essere letta come una piccola *captatio benevolentiae*: dal momento che ci troveremo,

momento che lo stato di salute di un Paese lo si misura sulla capacità del rientro e del virtuosismo fiscale, ossia sul tendenziale, sull'inversione della tendenza a sforare e a splafonare il debito sul prodotto interno lordo, ci si è dati degli obiettivi.

che ogni singola norma di un decreto‑legge deve rispondere ai requisiti costituzionali di straordinaria necessità ed urgenza. Adesso ditemi

di straordinarietà ed urgenza; a meno che non si dica che i pensionati in Italia muoiono di fame per cui è considerato straordinario ed urgente dare una risposta immediata alzando a livelli decorosi anche i minimi delle pensioni.

Ebbene, la Corte lo nega assolutamente e fissa un altro paletto, per la prima volta nella storia, dichiarando sostanzialmente che il Parlamento non può mai sanare la mancanza di presupposti costituzionali, altrimenti - ed è condivisibilissimo - si si scardinerebbe un principio costituzionale e il legislatore avrebbe addirittura la possibilità di alterare il riparto delle competenze, fissate in Costituzione, tra Parlamento e Governo. Questo non è possibile e lo ribadisce la Corte costituzionale. Il provvedimento che andiamo

nel nostro ordinamento, tre quarti delle norme che stiamo varando peccano di incostituzionalità. Forse l'unica, o una delle poche, che si salva sarebbe la famosa *probatio* diabolica invertita, in cui si consentirebbe a chi deve applicare indicatori di normalità economica di operare in termini di presunzione semplice, cioè invertendo l'ordine della prova nel caso dell'accertamento da parte dell'anagrafe da parte dell'anagrafe tributaria. Forse, visto che è già scaduto il termine per presentare le dichiarazioni, questa era l'unica norma costituzionale contenuta nel decreto.

alcune valutazioni sulle contraddizioni che tutto questo percorso mette palesemente sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda il metodo, questo Governo ci ha abituato a strozzare il dibattito parlamentare

il Governo, nel tentativo di approvare i provvedimenti, a porre il voto di fiducia. Non potete neanche negare ‑ questo lo dico per esperienza personale, ma questa valutazione non può essere confutata da alcun collega, anzi non potrebbe che essere condivisa dai colleghi della maggioranza - che quando, invece, esiste la possibilità di approfondire un argomento, di valutarlo, di sviscerarlo,

a proposito del provvedimento sull'*intramoenia*, con una scadenza del 31 luglio, provvedimento che ha ricevuto, dopo una lunga e approfondita discussione

il percorso della cosiddetta democrazia decidente, cioè quel percorso che permette di dedicare ai provvedimenti un certo tempo di discussione per poi arrivare all'approvazione. Il metodo esiste, è percorribile, è dimostrato che è possibile il confronto e anche la convergenza su provvedimenti importanti, ma - torno a ripetere - in realtà il vero problema per cui ponete la fiducia

tanto è vero, come diceva prima il collega, che questo è un provvedimento che destina circa il 70-80 per cento dell'entità del tesoretto (che poi ancora non si è capito bene quale sia) in spesa corrente. Allora, di fronte a questi elementi,

l'anno scorso avete varato una manovra finanziaria mettendo le mani nelle tasche degli italiani in modo pesante e ne avete pagato, fortunatamente, perché gli italiani non sono sciocchi, le conseguenze attraverso un calo di consenso piuttosto consistente nei confronti di questo Governo. Ve ne siete accorti Ve ne siete accorti e avete pensato di utilizzare il tesoretto nel tentativo di recuperare. Le forze che condizionano l'azione di questa maggioranza, però, hanno condizionato questo meccanismo di *marketing* politico e hanno portato ad un risultato diverso. Oggi la contraddizione che emerge, e che voglio mettere nell'ambito di questo dibattito in evidenza, è che, come dicevo, prima avete terrorizzato gli italiani in relazione alla situazione dei conti con la finanziaria dell'anno passato; poi, guarda caso, questi conti non erano così gravi, tanto è vero che c'è stato un gettito superiore che avete distribuito secondo una logica di

propone e annuncia che la prossima finanziaria sarà più leggera, sarà una finanziaria, si immagina, di circa 15 miliardi di euro. Bene, io mi sono permesso di fare alcuni conti e valutazioni di leggere alcune carte, perché poi è sufficiente fare queste cose, e mi sono accorto che i 15 miliardi euro sono un'altra di quelle *boutade* o un'altra di quelle scivolate alle quali andrà incontro questo Governo perché la realtà dei conti è ben diversa. Indìco solo una voce che vi farà sballare questi conti che è quella della spesa sanitaria e cito la fonte, cioè la relazione della Corte dei conti a Camera e Senato che, oltre a serie di valutazioni sul decreto «salvadebiti» sul disavanzo del 2005 (3 miliardi di euro), prende in esame i disavanzi del 2006, prende in esame i disavanzi del 2006, i disavanzi del 2007 e, siccome la spesa sanitaria ha un *trend* crescente, i disavanzi ipotetici del 2008. Ebbene, calcolate che agli ipotetici 15 miliardi di euro che dovrebbero costituire la manovra

è completa: avete aumentato le tasse, poi c'è stato un gettito superiore che avete usato per equilibri politici interni. Non contenti di questo dite che farete una manovra finanziaria che alleggerirà la pressione fiscale e, nello stesso tempo, i dati dimostrano che questo non avverrà: ne sono assolutamente convinto (e lo affermo oggi, non dico in attesa e in speranza, anche se essendo anch'io un cittadino italiano gradirei che alla fine la pressione fiscale diminuisse per il bene del Paese e le possibilità di crescita), perché le vostre capacità, che sono sul tavolo, mi fanno pensare che questo non avverrà. Di conseguenza, immagino e dico che ci troveremo nei prossimi mesi a discutere una manovra fiscale che sarà di circa 40 miliardi di euro. Questo significherà chiaramente che non diminuiranno le tasse e che probabilmente aumenteranno.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le considerazioni che seguono vogliono essere un invito formale rivolto al presidente Prodi e al suo Governo: abbiate il senso della responsabilità civile prima ancora che politica e istituzionale. Credo davvero non abbia più alcun senso continuare in una campagna di mistificazione da parte della sinistra sul lavoro svolto nei cinque anni di Governo Berlusconi. La legge finanziaria e il bilancio dello Stato per il 2007 contengono una mistificazione in ordine alla stima del totale delle entrate pubbliche, ancora oggi ufficialmente fissato a 703 miliardi di euro. Sulla base del gettito realizzato nel 2006 e dei dati presentati dal Governo nelle relazioni trimestrali, non si può parlare di "extragettito miracoloso" o "tesoretto", ma di "gettito nascosto" per circa 30 miliardi di euro. Il Governo deve dare risposte chiare, non muoversi mediante dissimulazioni e artifici contabili. Andiamo a vedere che cos'è il tesoretto. Il maggior gettito dovrebbe andare a ridurre *deficit* e debito pubblico, come per altro richiesto da tutti gli organismi internazionali, Unione Europea in testa. Il Presidente del Consiglio ha affermato: "In un anno abbiamo risanato i conti pubblici e il *deficit* 2007 sarà al 2,3 Peccato però che Prodi dimentica che il *deficit* pubblico è stato già al 2,3 per cento nel 2006, e non certo grazie al "tocco magico" del suo Governo. Quindi, dove sarebbe l'effetto Prodi-Visco? In realtà, poiché con la finanziaria 2007 il Governo ha aumentato di 35 miliardi la spesa pubblica ed ha aumentato le tasse più o meno dello stesso importo, ne consegue che il *deficit* di quest'anno è esattamente pari al *deficit* dello scorso anno. L'unica differenza, cioè il vero effetto Prodi-Visco, è un maggior peso fiscale dello Stato sui cittadini ed un maggior potere di spesa da parte dei Ministri, come sa bene anche il mio conterraneo sottosegretario Lettieri. Dopo gli allarmi dell'Unione Europea e del Fondo monetario internazionale sulla sostenibilità dei conti pubblici e del sistema previdenziale italiano, è arrivata per il Governo Prodi la doppia bocciatura della Banca d'Italia e della Corte dei conti. Presidente, le parole del governatore Draghi e del presidente della Corte dei conti sono di forte critica alla politica economica del Governo, tutta incentrata sulle tasse e su un indiscriminato aumento della spesa pubblica. Il giudizio di Draghi sul DPEF è particolarmente negativo in relazione alla favorevole congiuntura economica che "avrebbe consentito all'Italia di accelerare il riequilibrio dei conti in tempi brevi e non di rinviarlo al 2011». Il Governatore considera poi fuorviante parlare di "tesoretto" dinanzi a un debito pubblico come il nostro: "Queste risorse dovrebbero essere usate a riduzione del disavanzo e del debito perché altrimenti c'è il rischio di dover fare correzioni con un ciclo economico meno favorevole e comunque si sarebbe potuto ridurre la pressione fiscale anziché aumentare la spesa". Draghi è entrato con decisione anche nel dibattito sull' abolizione dello scalone pensionistico: «Per garantire nei prossimi anni delle pensioni adeguate a un numero crescente di persone bisogna aumentare l'età in cui si smette di lavorare». Draghi invita, quindi, il Governo a rivedere il sistema pensionistico tenendo conto del suo equilibrio finanziario per fare così un buon servizio ai giovani e alle future generazioni. Preoccupazione per l'alto livello della spesa pubblica è stata espressa anche dal Presidente della Corte dei conti, in «una lettura attenta delle stime di finanza pubblica per il 2007 sospinge ad un giudizio più allarmato sulle tendenze in atto, confermando tutte le preoccupazioni sulle difficoltà di controllo dei conti dello Stato». Per il presidente della Corte dei conti il cosiddetto tesoretto è ascrivibile soltanto «all'aumento delle entrate e della pressione fiscale», che è passata dal 40,6 al 42,4 E se il Governo vorrà rispettare gli impegni sottoscritti con Bruxelles, «anche la prossima legge finanziaria dovrà disporre una manovra in grado di ottenere risorse aggiuntive fino a un massimo di oltre 21 miliardi di euro». Quest'Assemblea, signor Presidente, il Paese, ha bisogno di risposte serie e coerenti, di opere e non di sterili personalismi polemici: né tantomeno dell'elargizione alla casta del centro-sinistra, al ceto di governo e di sottogoverno dei soldi prelevati sui sacrifici delle famiglie, degli imprenditori e dei professionisti di questo nostro Paese. Su questi interrogativi abbiamo bisogno di risposte vere e non fumose. Forza Italia dice no ad una odiosa tassazione. La Francia ha ripreso a correre abbattendo il carico fiscale e diminuendo la spesa pubblica inutile. Dobbiamo sostenere i lavoratori, le imprese, le famiglie, non vessarle con manovre finanziarie pesanti e che riducono la capacità di spesa e di risparmio di ognuno di noi. Il programma di lavoro del nostro passato Governo si basava su un assioma fondamentale: l'evoluzione del sistema economico legata indissolubilmente all'investimento pubblico e privato nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Il Governo Berlusconi ha elaborato e attuato nuovi programmi, di dimensione comunitaria e sovracomunitaria, i nuovi Corridoi transeuropei, la connessione del Corridoio 8 con la Puglia, le autostrade del mare, i grandi schemi idrici. Tutto ciò per modernizzare l'Italia e per renderla accessibile, per aumentare la libera e sicura circolazione di persone, di beni, merci e servizi; per rendere il nostro Mezzogiorno attraente per l'investimento produttivo, come ha già ricordato il senatore Gentile nel suo intervento. La nostra stella polare è stata l'operatività. L'idea di realizzare, giorno dopo giorno, una svolta epocale, dopo decenni di blocco di investimenti, di ritardi e di dispersione di risorse finanziarie e nelle opere pubbliche strategiche, nelle strade, nei porti, negli aeroporti, nelle ferrovie. Un ritardo che l'Italia e soprattutto il Mezzogiorno pagavano da decenni. Ci hanno attaccato violentemente, sulle piazze, sulle televisioni, sui giornali, denunciando fatti e persone di fronte alla magistratura. Hanno tentato di screditarci, dicendo che la legge obiettivo era stata un fallimento e che era stata un meccanismo inutile di spesa pubblica senza risultati. Oggi, il Governo Prodi, i ministri Di Pietro, Padoa-Schioppa, Bianchi e altri sono, loro malgrado, costretti a riconoscere che la legge obiettivo e il *master plan* delle opere sono stati l'operazione infrastrutturale più importante fatta in Italia nel dopoguerra: nonostante i radicalismi preistorici del ministro Pecoraro Scanio (che si è astenuto in Consiglio dei Ministri sull'allegato infrastrutturale) e della sinistra radicale (con la presidente Anna Donati che ha detto no all'allegato infrastrutturale), a testimonianza di una visione chiusa e cieca sulle potenzialità di sviluppo. Il DPEF presentato da Di Pietro e dal suo Governo, con l'astensione inspiegabile del Ministro dell'ambiente, è in sostanza una copia del Piano decennale delle opere presentato da Berlusconi, in cui viene presentato lo stato di avanzamento dei progetti e delle opere e nell'ambito del quale si articolano le temporalità progettuali e di realizzazione delle opere a seconda del reperimento delle risorse. Noi conosciamo la preoccupazione delle famiglie italiane, di quei professionisti e imprenditori che oggi devono pagare un'imposizione fiscale pesantissima e che costituisce un fattore di crisi di competitività del nostro Paese e del nostro Mezzogiorno. Chi può pensare di investire, di creare occupazione se le migliori risorse vengono convogliate, tramite un prelievo fiscale assolutamente non in linea con i Paesi dell'Unione Europea, a vantaggio di perversi meccanismi di devoluzione delle risorse per spese a favore di fondi di inefficienza della pubblica amministrazione? Come si pensa di incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro, di fronte a un prelievo fiscale così pesante? Noi siamo qui. Siamo qui per difendere il nostro territorio, il nostro Mezzogiorno. Non ci stancheremo di vigilare e di continuare a presentare un'alternativa di Governo seria, praticabile e concreta. La capacità di governo di Prodi e dei suoi referenti locali è stata misurata dagli italiani, che testimoniano ogni giorno la scarsità di risultati visibili e reali. Noi parlamentari di Forza Italia rimaniamo e rimarremo sempre a fianco dei nostri cittadini, ai quali vengono inopinatamente denegati diritti fondamentali tramite manovre di politica economica e finanziaria assolutamente prive di concretezza e lontane dalla domanda di benessere delle popolazioni, al di là della retorica e delle solite vuote strumentalizzazioni di una sinistra ormai prigioniera di se stessa, del dissenso interno e della crisi di consenso nel Paese. Per questi motivi annuncio il mio assoluto voto contrario a questo decreto.

esprimo un apprezzamento generale sul provvedimento nel suo complesso. In particolare, il mio apprezzamento va a quelle parti relative

È un provvedimento più volte richiesto e necessario, poiché tutti conosciamo le condizioni difficili in cui sono costretti a vivere milioni di anziani nel nostro Paese; in questi ultimi dieci anni, infatti, le pensioni hanno perso il 34 per cento di potere d'acquisto, per via del sistema di indicizzazione e del mancato aggancio alla dinamica salariale. Nondimeno, non mi posso esimere dal rilevare che l'aumento medio di 33 euro è da valutare come un primo segnale, piuttosto che come un reale e concreto intervento di sostegno a tale reddito. Il previsto utilizzo di una parte delle maggiori entrate nette rispetto al bilancio di previsione, il cosiddetto extragettito, per far fronte all'incremento dei trattamenti per i soggetti

stante l'esiguità dei redditi a tale titolo percepiti, vivono spesso in una condizione al di sotto della soglia di povertà, sia a livello individuale che familiare. In tal senso, non posso anche non apprezzare lo sforzo fatto dall'Esecutivo, oltre che con l'adozione delle summenzionate misure per l'anno in corso, anche mediante la previsione, per il prossimo anno, dell'istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un fondo finalizzato ad agevolare il riscatto a fini pensionistici della durata legale del corso laurea per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in regimi pensionistici diversi, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione in via esclusiva il regime pensionistico di calcolo contributivo, in modo da poter migliorare i i trattamenti previdenziali di un'ampia platea di soggetti, soprattutto i giovani, in quanto sono più direttamente interessati, da un lato, dal regime contributivo e, dall'altro, dai processi di modifica del mercato del lavoro e dalle nuove tipologie del cosiddetto lavoro flessibile, che in sostanza configurano rapporti di lavoro precario. Ultima, ma non ultima per significato e portata, è la disposizione che prevede l'applicazione di un meccanismo di indicizzazione del 100 per cento rispetto all'inflazione per tutte le pensioni fino a cinque volte il minimo; indicizzazione che ha costituito una bandiera di numerose battaglie condotte anche da me stesso in prima persona e dal mio partito ed inserita come impegno nel programma della maggioranza, che oggi trova finalmente riconoscimento. In conclusione, ritengo di poter valutare positivamente l'effetto redistributivo così raggiunto, ma sicuramente non posso ritenerlo sufficiente, perché - lo ribadisco - c'è nel nostro Paese la necessità che a questi interventi segua un'ulteriore coerente e penetrante azione del Governo, a partire dall'imminente e delicatissima manovra organica di riordino del sistema pensionistico e

A questo proposito voglio ricordare che sia in quest'Aula sia alla Camera l'approvazione del DPEF è stata accompagnata da precise indicazioni che ritengo debbano essere interpretate come vincolanti per il Governo; diversamente, penso si aprirà un difficilissimo periodo, in cui sarà davvero a rischio la tenuta di questa maggioranza. È per tale motivo che insisto perché si prosegua con una politica di redistribuzione sociale, in particolare attraverso misure che affrontino i problemi della precarietà del lavoro, che in particolare sia in grado, attraverso l'eliminazione della piaga del precariato, di ridare certezza

come è stato per le nostre generazioni e quelle precedenti, una vita ed una vecchiaia dignitose, invertendo così l'attuale situazione

Regolamento prevede che: «Un Senatore può mancare alle sedute dopo aver chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea». Per prassi consolidata, la richiesta non deve essere fatta solo da parte dell'interessato, ma può essere fatta dai Gruppi. Credo che il Regolamento dica qualcosa di diverso, ma diamo per buono questo. Quest'oggi sono in congedo cinque senatori a vita, la cui richiesta di congedo è stata formulata dal Gruppo e nessuna traccia vi è della volontà da parte degli interessati. Uno di questi, il presidente emerito Cossiga, con cui ho avuto il piacere d'interloquire poc'anzi, mi ha detto che non ha autorizzato nessuno a metterlo né in congedo né in missione. Credo che in questo momento stia contattando il Segretario generale per revocare questa richiesta da lui non autorizzata, ma a questo punto chiedo che lei trasmetta al Presidente, prima che si proceda al voto di fiducia di oggi, la richiesta di verificare che gli interessati, ovvero gli altri quattro, abbiano espresso e autorizzato la richiesta di congedo, perché diversamente siamo di fronte a un'usurpazione della volontà e dei diritti dei senatori.

sulla scia di quello che ha detto ora il collega Calderoli, c'è un aspetto che voglio ulteriormente sottolineare: è vero che quando un collega del Gruppo chiede di essere messo in missione, si rivolge al Presidente del Gruppo. Questo può Questo può valere per tutti i Gruppi, ma certamente non può valere per il Gruppo Misto, che per la sua conformazione è un Gruppo eterogeneo, dove confluiscono coloro che non hanno aderito a nessun altro Gruppo. Quindi, per quanto concerne la richiesta delle missioni da parte del Gruppo Misto deve essere fatta dal singolo senatore e non può essere fatta

non voglio mettere in dubbio questo; ma non può la Presidenza non prendere atto di quanto affermato dal senatore Calderoli, avendo egli incontrato uno di coloro che erano stati iscritti come in missione, non fare le dovute verifiche per vedere se anche gli altri quattro sono nella stessa condizione del senatore Cossiga. Aggiungo che va tolto dall'elenco dei senatori in missione sicuramente il senatore Cossiga, perché non posso pensare che la Presidenza - chiedo scusa per il bisticcio delle parole - pensi che il senatore Calderoli ha detto in Aula una cosa non vera.

Certamente la configurazione del Gruppo Misto è - come diceva il Presidente Matteoli - molto eterogenea, ma le idee di Ciampi non possono essere sostituite dalle idee di Turigliatto.

René de Chateaubriand diceva che l'ipocrisia è l'omaggio che il vizio rende alla virtù. Il voto di fiducia è un istituto previsto dalla Costituzione, è stato sempre utilizzato, in ogni tempo; indubbiamente deve essere fondato su solidi motivi, su ragioni riconducibili alla *ratio* della Costituzione. Il decreto‑legge è un provvedimento di urgenza; non può l'urgenza essere sostituita da altro criterio di valutazione. Orbene, guardando questo provvedimento - ripeto osservazioni e obiezioni che sono state avanzate da rappresentanti delle opposizioni - esso innanzitutto non ha ha i requisiti che ne giustificano l'adozione e, soprattutto, la sua introduzione in Parlamento;

senza pregiudiziali immediate, di risultati immediati, si chiede quale sia la bussola che sta usando questo Governo, quale percorsi esso si stia dando; infatti, tutti gli atti di politica economica e finanziaria di questo Governo, dal DPEF alla legge finanziaria dello scorso anno, ad oggi, sembrano procedere lungo uno zig-zag che non rende comprensibile il traguardo. Si potrebbe dire, dopo questo provvedimento, che il Governo, pur di tenere la propria maggioranza - è un'osservazione già fatta - abbia dispensato alcune risorse a seconda delle varie richieste. E c'è da chiedersi perché oggi il Governo fa questa scelta, perché se fossimo alla vigilia delle elezioni, essa sarebbe anche comprensibile se non giustificabile. Non dovremmo essere alla vigilia delle elezioni, comunque, non dovremmo votare questo autunno. Allora, la questione diventa ancora più inquietante: un Governo che si annuncia come un Governo delle riforme, come il Governo che si cimenterà con il tema impegnativo del debito pubblico, appena consegue - ammesso che sia effetto e risultato della legge finanziaria dello scorso anno - un qualche risultato, pensa subito a disperderlo, invece che concentrare quel risultato nella finalità principale, che dovrebbe essere il risanamento e il taglio del debito pubblico. C'è una notizia di ieri che dovrebbe fare riflettere tutti, Governo, maggioranza; e certamente rifletta l'opposizione che trova una ragione di rafforzamento delle proprie ragioni oppositorie. Gli istituti di *rating* hanno valutato verso la tripla A i buoni del Tesoro provinciale, sale lo *spread* con i titoli tedeschi, il che significa che il costo del debito pubblico nei prossimi cinque mesi avrà un'impennata. Avremo non soltanto un incremento del debito pubblico, già molto elevato, ma anche un incremento del costo del debito pubblico. Orbene, una corretta manovra di risanamento finanziario è proprio su questo punto che deve far leva. I colleghi della sinistra cosiddetta radicale hanno posto sempre in questi mesi il tema dell'equità e vi sono argomenti da loro addotti che trovano corrispondenza anche negli argomenti delle opposizioni;

negli ultimi dieci anni hanno subito, hanno percorso una curva discendente: potremmo certamente dire che negli ultimi dieci anni larga parte degli italiani è diventata più povera. povera. È un dato che non si oppone a questa o quella maggioranza: è una constatazione che dimostra la incapacità, in questa lunga stagione, in queste ultime tre legislature che partono dal 1992, di affrontare quel tema del debito pubblico che è stato l'oggetto di una demonizzazione per la quale nel Paese si è aperto un processo politico,

a dire quelle per le quali una politica della Banca d'Italia ha imposto un rapporto lira-marco, che ha indotto l'incremento del debito pubblico oltre ogni dimensione prevedibile. Quello stesso errore, allora attribuibile alla politica monetaria della Banca d'Italia, viene ripetuto oggi per l'incapacità di affrontare e dominare il problema del debito pubblico e del relativo costo e, ancor di più, e, ancor di più, di un costo che viene pagato non già sul mercato nazionale in favore di *rentier*, di redditieri nazionali, ma sul mercato mondiale. I colleghi della sinistra radicale pongono i temi delle nuove povertà e del contrasto agli evasori (sull'uno e sull'altro argomento siamo perfettamente d'accordo), ma non pongono il tema del costo del debito pubblico che va a vantaggio soltanto del sistema finanziario mondiale, del quale si deve prendere atto non con parole di demonizzazione, ma con la capacità di intervenire sulle proprie condizioni, per tagliare il debito pubblico.

sul controllo di questa spesa pubblica che invece sembra regolarmente impazzita ‑ che ogni sopravvenienza attiva del sistema tributario venisse tutta concentrata in questa stagione, vale a dire alla vigilia dell'estate, nel taglio del debito pubblico, con una posizione attendista anche nei confronti dell'autunno. Il quadro dei dati fondamentali e della situazione economica, innanzitutto internazionale e poi nazionale, non confortano nel senso di una previsione di un incremento del PIL che sia la base ad un incremento del gettito tributario come quello stimato dal Governo, che ritiene di adottare una procedura che in altri tempi dispregiativamente si chiamava dorotea (io dei dorotei invece ho grandissimo rispetto), per la quale il consenso veniva acquistato quotidianamente o settimanalmente: una procedura che ha rappresentato la ragione della crisi di una stagione, di un assetto politico e che viene oggi rinnovata. La domanda è dunque la seguente: dove ci vuol portare questo Governo? Senza fare il profeta di sciagure (nessuno lo vuol fare), è fin troppo ovvio che i dati dell'incertezza potrebbero indurre lo stesso Governo, in autunno, ad un prelievo fiscale in contraddizione con la linea ulteriore che si sta seguendo, seguendo, sottoponendo il Paese ad uno *stress* in una fase in cui, invece, va sostenuta la ripresa produttiva, va sostenuta la capacità del Paese di reagire ai problemi e di di impostare - e questa dimensione è totalmente assente in questo Governo - la soluzione ai problemi del Paese. Guardando questo decreto, c'è un punto che è elemento che permette una valutazione, se non un giudizio politico *tranchant* definitivo: si introducono norme di finanza eccezionale per le Province contigue con le Regioni a Statuto speciale. Una cosa così aberrante con un decreto‑legge non poteva essere immaginata se non da chi ha l'esigenza di fronteggiare le mille domande del Paese, mediate, rappresentate e riflesse in questa maggioranza composita,

All'indomani della guerra, quando era aperto il problema della ricostruzione del Paese, De Gasperi con Vanoni - che non era né meridionale, né siciliano, siciliano, ma veniva da una regione del Nord - impose una scelta al Paese, cioè che accanto alla ricostruzione partisse lo sviluppo del Mezzogiorno. Orbene, oggi questo Governo non è capace di una proposta di disegno nazionale. Questo Governo, questa maggioranza, prende i voti nelle Regioni del Sud, che controlla politicamente, perché il governo di tutte le Regioni, ad eccezione della Sicilia, è nelle mani del centro‑sinistra; però, perde nel Centro-Nord e insegue allora le Province limitrofe alle Regioni a Statuto speciale,

chi ricorda le cose di questo Paese sa che in nessuna stagione il dialogo tra maggioranza e opposizione è stato chiuso e il voto di fiducia è stato il ricorso all'estrema necessità

Onorevoli senatori, basterebbe rileggere attentamente le dichiarazioni del senatore Morando per trovare tutti gli argomenti

che un Gruppo come l'UDC rinnova la propria posizione all'interno dello schieramento di opposizione, contrasta questo indirizzo del Governo, espone la propria posizione davanti al Paese e non può non far rilevare l'estremo insuccesso del tentativo del Partito democratico. Oggi nessuno si sottrae, in Italia, non dico alla suggestione, ma all'argomentazione per la quale occorra una evoluzione del sistema politico. Siamo in una stagione postideologica, probabilmente, anzi sicuramente è impossibile pensare che in Italia, in ragione delle diverse tradizioni culturali, ma anche della dominanza di interessi regionali, vi siano soltanto due partiti. Che a sinistra si stia formando il partito democratico potrebbe essere considerata, anche da parte di chi sta dall'altra parte, una ragione alla quale essere molto attenti e rispetto alla quale atteggiarsi emulativamente, guidando quindi un processo di riaggregazione ordinata, secondo un pensiero politico. Invece, questo non sta avvenendo perché il partito democratico, che è la base essenziale di questo Governo, si è annunciato come il partito delle riforme. Anzi,

che in Italia mi sembra non vi sia e che, comunque, non c'è nel centro-destra, perché quest'ultimo avverte le stesse ragioni, gli stessi stimoli e le stesse necessità

il partito democratico dimostra di non avere la forza di percorrere questo sentiero perché è sottoposto alla fortissima tensione e alla fortissima concorrenza della sinistra radicale. Orbene, è questa difficoltà che si rovescia, ancor prima che sulla situazione politica del Paese, sulla condizione della maggioranza. Ebbene, sono queste le ragioni per le quali da parte nostra il dovere della opposizione è indefettibile.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, con l'apposizione della questione di fiducia anche su questo provvedimento assistiamo ad un ennesimo esproprio della facoltà del Parlamento di espletare la funzione legislativa assegnatagli dall'articolo 70 della Costituzione. Si combina l'ennesimo pasticcio,

disponibili 1.952 milioni di euro per vari Ministeri e varie necessità. Ora, sappiamo da tempo - lo disse il ministro dell'interno Amato all'inizio di luglio dell'anno scorso - che una delle emergenze e delle maggiori necessità del nostro Paese è quella di tutelare la sicurezza.

Qualche giorno dopo il Governo approvò il decreto Bersani che tagliò 80 milioni di euro all'Arma dei carabinieri e 200 milioni di euro alla Polizia. in grande coerenza con quanto uno dei più importanti Ministri aveva evidenziato.

per i servizi di accoglienza a favore degli stranieri e 779.000 euro per l'assistenza economica e sanitaria sempre a favore degli stranieri. Si tratta di un chiaro esempio delle priorità che ha osservato questo Governo. Governo allora si è appropriato, ormai direi in tutta la legislatura, della funzione legislativa che la Costituzione assegna al Parlamento.

A seguito di mie interrogazioni, più volte sollecitate, sei mesi dopo ci è stato detto che effettivamente il Consiglio dei Ministri l'aveva autorizzata: sicuramente è vero, ma è strano che nella conferenza stampa tenutasi qualche minuto dopo il depositario degli atti del Consiglio dei ministri abbia negato l'autorizzazione a porre la fiducia. E così, una bella serie di norme, di finte liberalizzazioni e vere tasse, sono state poste con il decreto Bersani.

per leggiucchiare, più che altro per soppesare, perché non si è potuto fare molto altro, nel quale vi sono stati i pasticci più inusitati. Ad esempio, fatto del tutto veniale, c'era un provvedimento, peraltro non negativo, riportato due volte.

che avessero regolarizzato secondo determinate modalità eventuali dipendenti non regolari fossero esentati per un anno dai controlli relativi alla sicurezza sul lavoro: un'altra bella ciliegina messa su questa ricchissima finanziaria.

più importante che segue (visto che il DPEF è risultato essere una presa in giro, perché non contiene le cifre più importanti), l'attuale decreto-legge. Per non sbagliarsi,

In nome di tali prerogative, la coalizione, nell'unico successo ottenuto nel corso di questi mesi di Governo, è riuscita a convincere un numero sufficiente di italiani a votare contro la riforma che la Casa delle Libertà aveva approvato nella scorsa legislatura. Il Governo ci è riuscito convincendoli che quella riforma sminuiva il ruolo del Parlamento, cosa assolutamente non vera, salvo poi espropriare in ogni modo il Parlamento dalle sue prerogative. Non ci sono soltanto i voti di fiducia, ma anche i decreti‑legge convertiti in fretta e furia, dove, di fatto, il Parlamento non può fare nulla. Ci sono inoltre le leggi delega, con cui, con pochi commi spesso confusi, si delega il Governo a legiferare su un vasto settore. Per fortuna, il Governo non riuscirà a farlo nella maggioranza dei casi per le sue divisioni interne, ma il danno resta,

alla base di questo anno di attività politica, portata avanti dal Governo e dalla maggioranza, che riguarda sia il metodo che il merito dell'attività di Governo. stato caratterizzato da un uso sproporzionato e da un abuso del ricorso allo strumento della fiducia, che ha finito con il mortificare le prerogative proprie del Parlamento. Con quella di oggi, colleghi, siamo, alla ventunesima richiesta di fiducia. stato caratterizzato da una forte irresponsabilità che questo Governo ha fatto registrare nei confronti delle attese del Paese e, soprattutto, delle giovani generazioni. delle giovani generazioni. Ritengo che questa sia una delle manovre più irresponsabili che un Governo abbia mai varato, soprattutto nei confronti delle future generazioni, sulle quali si scaricheranno gli effetti del provvedimento in approvazione.

Cosa significa infatti extragettito, tesoretto da porre a base di una manovra distributiva per un Paese che presenta un *deficit* che viaggia fra il 2 e il 3 per cento e che presenta un debito pubblico prossimo al 105‑106 Per un Paese come questo non esiste extragettito o tesoretto da porre a base di qualsiasi manovra distributiva; tanto più quando si tratta di una manovra di chiaro stampo elettorale, quale quella che emerge dagli interventi di spesa messi in campo dalla manovra stessa. Tali interventi attengono alle misure più disparate, e non sto qui a richiamarle per economia di tempo,

in relazione alle opere messe in campo; l'extragettito non è disponibile per manovre distributive. Questo non lo stiamo dicendo solo noi: lo dicono e l'hanno detto le più significative istituzioni economiche europee; l'ha detto e continua a dirlo il governatore della Banca d'Italia Draghi. Allora, se l'extragettito non esiste, se il tesoretto non esiste, se questa risorsa non può essere disponibile per nessuna manovra in un Paese come il nostro, con i dati che si porta dietro, è necessario, secondo me, indagare su quale sia stato il ragionamento che ha portato avanti il Governo per mettere in campo una manovra distributiva di 7 miliardi di euro. Penso che questo Governo abbia ragionato in un modo

licenziata in un momento elettorale, aveva guardato agli interessi del Paese. A fronte di questo extragettito e di queste maggiori entrate, l'esercizio di bilancio può essere chiuso con un disavanzo netto pari al 2,1 Dato, però, che le previsioni portavano ad un indebitamento netto del 2,5 per cento, allora è possibile effettuare una manovra distributiva pari allo 0,4 per

Per la prima volta si assiste in Europa ad una manovra tesa ad aumentare il disavanzo. È un *record*, ma non è l'unico che detiene il nostro Paese, atteso che per la prima volta in un Paese europeo si è proceduto, con la controriforma delle pensioni,

se va bene, 78-80 miliardi l'anno. Si interviene correndo anche il rischio che la responsabilità dei futuri aumenti dei tassi d'interesse da parte della Banca Centrale Europea finirà per essere addossata all'Italia, all'Italia, che ha mantenuto un debito pubblico così elevato per così lungo tempo. Allo stesso modo all'Italia potrà essere addebitato il fatto che a causa di un debito pubblico così elevato il rapporto di cambio euro-dollaro possa divenire molto sfavorevole alle nostre esportazioni e a quelle europee. Si tratta di una manovra poco responsabile, perché tra l'altro, a fronte di voci di spesa strutturali, che si ripetono negli anni, non vi è certezza relativa alla valenza strutturale delle maggiori entrate. Non siamo, cioè, oggi sicuri che l'extragettito si manifesterà anche negli anni futuri, con conseguente spesa non coperta in futuro. Ciò comporterà, tanto per cambiare, un inasprimento della pressione fiscale. Come stride, come contrasta, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, questa manovra e il suo contenuto con quanto dichiarato da Veltroni a margine del dibattito conseguente alla sua candidatura a capo del nascente Partito Democratico,

per il Governo e la difesa degli interessi della società in essere; il centro-sinistra, invece, è una coalizione che si propone per il Governo e la difesa degli interessi delle generazioni future. Per quella che è stata la storia del centro-destra e del centro-sinistra negli ultimi dieci anni, per quella che è stata la politica portata avanti dal Governo di centro-sinistra nell'ultimo anno e per quello che è il contenuto del provvedimento in esame, possiamo tranquillamente affermare che mai definizione si rivelò tanto fallace. tanto fallace. A parte le dichiarazioni di Veltroni, un minimo di attenzione nei confronti delle giovani generazioni ce lo saremmo aspettato, anche per fare giustizia dell'onere che andrà a gravare sui giovani a causa della controriforma messa in campo dal Governo in materia previdenziale per superare lo scalone. Mi riferisco agli oneri contributivi aggiuntivi che andranno a gravare sulle categorie più deboli dei lavoratori, come i giovani lavoratori e i parasubordinati, che vedranno aumentare fino a tre punti l'aliquota contributiva per raccogliere i 4,4 miliardi necessari per far fronte, parzialmente, all'aumento di spesa che l'annullamento dello scalone comporta, circa 10 miliardi in 10 anni. Aumento di aliquota contributiva che avrà gravi ripercussioni sui livelli occupazionali e sulla qualità del lavoro. Siamo convinti che aumenterà il lavoro sommerso perché si tratta di un provvedimento assunto senza alcun riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro. Presidente, signor Sottosegretario, anche perché annunciato, ci saremmo aspettati finalmente che questo Governo, atteso il momento congiunturale favorevole, ponesse mano finalmente ad una revisione degli ammortizzatori sociali. È un provvedimento che il mondo del lavoro attende da fin troppo tempo, dal 1997, quando fu varato quell'insieme di norme che passarono poi sotto il nome di pacchetto Treu e che introdussero per la prima volta il concetto di lavoro interinale e di lavoro flessibile. Se si accantona, se si mette da parte la velleità, tutta ideologica, di procedere ad una controriforma della legge Biagi, attesi i risultati positivi prodotti in materia occupazionale, bisogna prendere atto che quella riforma va completata per ciò che attiene il regime delle tutele; nuovo regime di tutele che vadano a proteggere il lavoratore non solo e non tanto nel rapporto di lavoro ma che accompagnino e proteggano lo stesso lavoratore nel mercato del lavoro, tutele che costano, riforme che costano. Si poteva cogliere l'occasione dell'extragettito, se proprio non doveva essere utilizzato per opere di risanamento, per avviare una riforma che è l'unica possibile capace di contrastare la precarietà, l'unica riforma possibile che potrà fare in modo che la flessibilità, necessaria per un mondo produttivo in evoluzione, non si trasformi in precarietà. ce la aspettavamo per il Mezzogiorno d'Italia, convinti come siamo che la sfida della competitività questo Paese la vincerà solo e soltanto se sarà in grado di liberare le risorse potenziali del Mezzogiorno d'Italia, risorse potenziali che per essere

ponte per i Paesi del Mediterraneo. Tutto questo non c'è, non si riscontra in questo provvedimento, ed ecco perché noi voteremo contro la fiducia a questo Governo. Ci auguriamo settembre e ottobre siano la stagione della fine di questo Governo per il Paese e per i giovani italiani. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, oggi ci troviamo a discutere del cosiddetto tesoretto. Il Governo ci ha spiegato che si tratterebbe dell'extragettito maturato nei primi mesi del 2007. Allora la prima domanda che mi sento di porre è la seguente: esiste davvero questo extragettito? Noi pensiamo di no e, nel nostro giudizio, siamo confortati anche dal parere espresso pochi giorni fa dal governatore della Banca d'Italia Draghi che, in audizione davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, ha testualmente affermato che non esiste un tesoretto da spendere, che la parola tesoretto è fuorviante e che il miglioramento delle entrate, che sono derivate dalle maggiori imposte che gli italiani hanno pagato per effetto dell'ultima finanziaria, avrebbe dovuto essere utilizzato per diminuire il *deficit* di bilancio, per migliorare i saldi contabili, perché il *deficit* pubblico, contrariamente a quello che dice il presidente Prodi, è tutt'altro che sotto controllo. Ed infatti anche il commissario europeo Almunia, la Corte dei conti e il Fondo monetario internazionale continuano ad esprimere riserve e critiche nei confronti delle vostre scelte di politica economica. L'impegno al contenimento del *deficit* di bilancio era previsto dalla vostra ultima legge finanziaria per il 2007 che stabiliva che eventuali fondi in più, che fossero risultati dalle maggiori entrate fiscali maturate nel corso del 2007, dovevano essere utilizzati per il ripianamento del debito. come avevate sempre affermato, la priorità per il 2007 era il risanamento dei conti, e per questo avete imposto sacrifici a tutti i contribuenti italiani, perché ora dilapidate il risultato di questo sforzo collettivo in una miriade di interventi a pioggia, di marchette politiche, che non costituiscono una vera politica economica, ma solo clientela e sperpero di risorse pubbliche? Ricordo alcune di queste i 700 milioni in più di spesa, che sono stati lasciati ai Ministeri; i fondi per la cinematografia che forse servono per aiutare la campagna elettorale all'interno del Partito Democratico di Walter Veltroni; ulteriori 80 milioni per lo scandalo delle immondizie napoletane. La riprova di quanto sto affermando la troviamo nel disposto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge in esame, che dispone il disaccantonamento di somme previste come risparmio della legge finanziaria per il 2007. Quindi, prima con la finanziaria avete bloccato quelle spese, affermando che si trattava di risparmi finanziari, ma ora, in totale contraddizione con tale lodevole intenzione, a pochi mesi di distanza consentite ai Ministri di spendere quelle stesse somme. Ma di che risparmio si trattava allora? E' questa la prova provata che l'ultima finanziaria è stata tutta un errore. Non era necessario imporre nuove tasse e punire gli italiani per risanare il *deficit* lasciato dal Governo precedente come, mentendo agli italiani, avevate detto, ma invece quelle nuove tasse erano necessarie solo per alimentare la voragine della spesa pubblica di parte corrente, le clientele dei Ministri, come in concreto oggi dimostrate di fare. Anche la Francia, come il nostro Paese, ha difficoltà a rispettare gli impegni presi in sede europea di eliminare il *deficit* di bilancio: anche Sarkozy, come Prodi, si è recato a Bruxelles invocando una rimodulazione del piano di rientro del *deficit*, ma guarda caso ha trovato, al contrario di Prodi, comprensione delle autorità europee. Sarkozy, infatti, appena rientrato da Bruxelles, si è recato all'Assemblea Nazionale e ha varato due poderose riforme economiche: la prima, la defiscalizzazione totale del lavoro straordinario; la seconda, la totale flessibilità per tutti i neoassunti nelle imprese. Queste sono vere liberalizzazioni, altro che le patacche, spacciate per liberalizzazioni, che ci ha propinato il ministro Bersani. il ministro Bersani. Con questa robusta iniezione di energie positive la Francia dimostra di avere le carte in regola per avviare un *trend* economico di crescita, con il quale finanziare la riduzione del *deficit*. Voi invece che fate? In controtendenza con tutta l'Europa, decidete di modificare lo scalone Maroni e di abbassare l'età minima per andare in pensione, che tra l'altro era già la più bassa di tutta Europa. E come finanziate questo costo? Aumentando i contributi previdenziali sui lavoratori atipici, quindi su giovani e precari, proprio le categorie che, a parole, dichiarate di voler tutelare. Tutto il mondo economico internazionale assiste sconcertato a queste vostre insensate scelte di politica economica. In genere è tipico che all'inizio di legislatura i Governi attuino politiche di rigore e di risanamento dei conti, e solo negli ultimi anni della legislatura, in vista delle elezioni, diano corso a politiche clientelari per recuperare consenso. Voi, al contrario, dopo un solo anno di Governo, date immediatamente corso alla spesa facile. E' del tutto evidente che siete consapevoli che proprio così non potete andare avanti, che la maggioranza al suo interno è lacerata. Troppe cose vi dividono, dalla politica estera alla politica economica: le elezioni incombono, probabilmente già la prossima primavera. E' per questo che per l'ennesima volta vi negheremo la fiducia, che avete già perso nel Paese, come risulta ormai da tutti i sondaggi e dall'analisi di tutti i più autorevoli commentatori politici. *(Applausi

la Thatcher, di fronte a chi la ammoniva sulle conseguenze che l'ondata mercatista avrebbe prodotto sulla società, disse: «La società non esiste». Invece la società esiste, ed è sempre più terribilmente diseguale; si è sgranata una condizione sociale e la società è sempre più terribilmente diseguale diseguale di fronte alla fase che chiamiamo globalizzazione, di fronte ad un capitale spesso senza capitali. Eppure nel nostro Paese la produttività del lavoro nei settori delle costruzioni e delle manifatture è la più alta d'Europa, con un costo del lavoro che è il più basso per unità di prodotto, che poi è quello che conta nella competitività. Esiste la società nella condizione di tanti anziani dopo una vita di lavoro; basta vedere i dati INPS sui rendimenti della nostre pensioni. Esiste la società nella condizione di precarietà dei giovani; giovani generazioni che stanno peggio dei loro padri, e spesso dei loro nonni, in una condizione di precarietà e flessibilità. Esiste la società,

appunto della disoccupazione agricola. Esiste così tanto la società e la sua condizione materiale che ieri, insieme al Presidente della Camera, il Presidente del Senato (è oggi su tutti

che segnano la condizione sociale nel nostro Paese. Secondo dati del Governo, il 63 per cento delle aziende sottoposte a controllo è risultato non in regola

Oggi, con questo provvedimento, viene proposta una manovra che parla di redistribuzione delle risorse, di un aumento delle pensioni minime,

genere è appunto penalizzata - che con l'ipotesi dell'aumento a 64 anni vengono penalizzate ulteriormente le donne, che hanno una vita lavorativa e pensionistica differente, come indicano le statistiche, che qui non cito, e una diversa età pensionabile. Avremmo preferito una differenziazione anche di quel

Non si può non ricordare che nella Commissione competente giacciono disegni di legge per la tutela delle bambine e dei bambini, per il sostegno alle famiglie più disagiate

rispettate le conversioni sulla via di Damasco, ma il Governo non ha operato come Robin Hood nella foresta di Sherwood, anche se consiglierei al Governo di avere più propensione ad essere Robin Hood e a sconfiggere quell'idea che, come abbiamo visto,

rendimento della sua capacità. Per tali ragioni dicemmo, anche prevedendo questi ragionamenti, che la finanziaria passata avrebbe potuto essere più leggera.

Quei lavoratori denunciavano che il vice presidente della Confindustria Tognana, che ha un ruolo di rappresentanza generale del sistema di imprese nel nostro Paese, ha chiuso a Manfredonia una fabbrica

di uomini e donne che vivono del proprio lavoro, lottando per modificare e migliorare le loro condizioni e le condizioni di quel lavoro. Attraverso questa via si cerca di creare nuove e più avanzate condizioni per la loro vita e per tutta la

Ho apprezzato i richiami ai livelli di democrazia nella maggioranza che ci vengono dall'opposizione. Non c'è nessuna costrizione a votare questa fiducia, ma anzi una convinzione per la natura e per quello che parla alla società nel nostro Paese. È certo però e lo dico al Governo - che questo voto segna un passaggio di fase che sta appunto nelle condizioni materiali della società di cui parliamo.

dicevo prima - se, attraverso la politica, nota un miglioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro. Solo così la politica torna ad essere un fatto di massa, l'azione di governo si peggiora quella condizione di vita, il distacco tra politica, società e condizioni materiali senz'altro aumenterà. Per questo noi abbiamo avanzato alcune critiche. É stato qui ricordato che si diminuisce l'età pensionabile. Noi parliamo di condizioni concrete e condizioni materiali di vita; parliamo di quei 1.300 morti sul lavoro, non dati da sbadataggine, ma dalle condizioni dell'organizzazione del lavoro e dai rapporti capitalistici di produzione; sono sono vittime del sistema, è quella condizione, è quella umanità che appunto prima ricordavo. Quel protocollo che parla di pensioni e *welfare* va cambiato. Parafrasando quello che diceva il sindacalista Benvenuto davanti alla FIAT, dico che o cambia il protocollo o il protocollo cambia, perché quello, in qualche caso, aumenta l'età pensionabile, anche con riferimento alla condizione di precarietà di tanti giovani. Il Governo sa che il nostro sì è sì e il nostro no è no. Oggi con lealtà e convinzione condividiamo il segno del provvedimento in discussione e la fiducia che viene viene richiesta. Domani deve aprirsi un confronto nella maggioranza e nel Governo per modificare quel protocollo. Lo dobbiamo a quella umanità di cui parlavo prima, che non è un'altra umanità, ma è la nostra.

questo provvedimento è particolarmente emblematico della politica del Governo con riferimento al rapporto che essa assume tra crescita e coesione sociale. Potremmo dire, analizzandolo e combinandolo con il recente protocollo offerto alla firma delle parti sociali, che esso si pone in coerenza con la politica enunciata dal *leader* designato del Partito Democratico. Democratico. Quando nei giorni scorsi, nel vivo della complessa trattativa sul sistema previdenziale, ho visto un articolo di Veltroni sulla prima pagina del quotidiano «la Repubblica», ho per un attimo pensato ‑ forse temuto potesse contenere un'indicazione forte e chiara sulle necessarie opzioni di un nuovo modello sociale per l'Italia. Già la lunghezza del pezzo mi fece intuire ciò che leggendolo avrei appreso: Veltroni, come tutta l'Unione e il suo Governo, non sceglie, ma somma tutte le possibilità politiche sociali, con il risultato di non conferire ad esse la forza della spinta per un nuovo modello di società, la qualità della sostenibilità finanziaria nel medio e lungo periodo, il vantaggio della compatibilità con i doverosi obiettivi di riduzione della pressione fiscale e contributiva. Il Governo, infatti, non sceglie una più moderna composizione della spesa sociale in modo che questa sia riorientata dalle vecchie logiche assistenziali alla promozione di una società attiva, ovvero di una società che valorizza il proprio capitale umano ed è perciò insieme più inclusiva e più competitiva. Esso non ha il coraggio di produrre, e nemmeno di confermare, riforme utili a stimolare un modello di *welfare* *community* e a spostare significative risorse pubbliche dalle vecchie pratiche della protezione passiva a quella tutela attiva che si realizza attraverso il sostegno alla famiglia e alla capacità di procreazione, un rinnovato sistema educativo e formativo, la borsa del lavoro ed una convinta promozione della pluralità dei servizi per l'impiego, la rivalutazione del lavoro attraverso retribuzioni e trattamenti fiscali che premino il merito e l'impegno professionale, il ridisegno di forme responsabili di tutela della salute, un sistema previdenziale fondato sull'equilibrio tra prestazioni e contribuzioni come sul preveggente accantonamento di risorse complementari. Il decreto ed il protocollo - che invero pochi sembrano davvero disponibili a firmare per intero - cumulano invece vecchie e nuove impostazioni, con il risultato di un rilevante incremento della spesa corrente, di una inevitabile ed ulteriore lievitazione della pressione fiscale e contributiva nel Paese, ove, non a caso, gli alti livelli del prelievo si coniugano con la straordinaria dimensione del lavoro sommerso e, ancora, di segnali ambigui e contraddittori in relazione all'obiettivo di una società attiva. In particolare, ad esempio, la spesa aggiuntiva per i pensionati disagiati si collega solo in parte a ciò che il Governo Berlusconi aveva lodevolmente avviato, ovvero l'idea di una sorta di reddito minimo garantito agli anziani che non sono in età di lavoro, tenendo conto non solo del reddito individuale, ma anche di quello del nucleo familiare, necessario presupposto per un intervento straordinario dello Stato. Con questo approccio voi mescolate un intervento altrettanto assistenziale, perché non sostenuto da versamenti contributivi, ma a questi proporzionato, che è rivolto a sostenere il reddito di pensionati che ricevono una modesta prestazione previdenziale, senza tenere conto del reddito familiare.

per cento dell'incremento di queste pensioni andrà - secondo una simulazione scientifica dello stesso Baldini che, utilizzando il campione rappresentativo delle famiglie italiane, determina il noto indice di Gini sulla distribuzione del reddito - a favore di famiglie appartenenti alle fasce di reddito più alte. Lo stesso sostegno ai giovani, pur condivisibile quando agevola la totalizzazione da noi avviata dei contributi contributi o il recupero del periodo di laurea o quando riprende la nostra idea di un fondo per garantire l'assunzione di debiti bancari, lo diventa meno quando ipotizza una facile e deresponsabilizzante copertura previdenziale delle interruzioni tra le prime esperienze lavorative o quando, più in generale, scarica sulle giovani generazioni tutto l'onere di un sistema previdenziale generoso in termini di età di ritiro dal lavoro. L'impegno per un tasso di sostituzione del 60 per cento dell'ultimo reddito è poi particolarmente ridicolo perché è irrealizzabile o garantito da un forte impegno della fiscalità generale e, perciò, a carico degli stessi giovani che ne dovrebbero beneficiare. Non è un caso, infine, che in questo provvedimento, dedicato a bruciare con tempestività le maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007, ritornino gli studi di settore e il nodo della retroattività dei nuovi indicatori di normalità che li hanno unilateralmente modificati. Con la usuale ambiguità, il Governo accoglie parte delle richieste avanzate da noi e da componenti della stessa maggioranza, lasciando intendere che nel caso di accertamento non vi sarà inversione dell'onere della prova. La fiducia impedisce di esaminare il nostro emendamento, che avrebbe in radice eliminato ogni possibilità di applicazione retroattiva, o di approvare l'ordine del giorno della collega Thaler Ausserhofer, per una più certa interpretazione del testo. Nel frattempo, i professionisti che assistono gli operatori nella dichiarazione dei redditi consigliano di non tener conto dei nuovi indicatori ai quali voi assegnate invece un definito gettito aggiuntivo. La sintesi è che avete, ancora una volta, scoraggiato lo sviluppo della leale collaborazione fra fisco e contribuente, facendo regredire il percorso virtuoso che si era avviato, con quei risultati che hanno consentito proprio questo provvedimento. Ed è anche per questa ragione che le spese che qui decidete non saranno per nulla sostenibili.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il provvedimento sul quale il Governo ci chiede di esprimere la fiducia è pieno di buone notizie per gli italiani. Contiene buone notizie per oltre tre milioni di pensionati al minimo, per il regime previdenziale dei giovani, per le imprese con lo sblocco della riduzione del costo del lavoro di tre punti deciso in finanziaria, con la reintroduzione della deducibilità dei costi per le auto aziendali oltre al rimborso IVA auto e allo sblocco di incentivi e misure per fronteggiare le crisi d'impresa, per gli artigiani, i commercianti e i professionisti con la definizione di un nuovo e importante principio giuridico connesso all'attuazione degli studi di settore ovvero l'affermazione della non automaticità degli accertamenti e della natura di presunzione semplice degli indicatori di normalità, norme queste - come è noto - definite presso la Commissione finanze del Senato e recepite durante l'*iter* di conversione del decreto-legge alla Camera dei deputati. Misure importanti riguardano i Comuni (con l'autorizzazione - seppur parziale ad utilizzare gli avanzi di amministrazione), le infrastrutture (con lo sblocco parziale del fondo TFR, ulteriori trasferimenti a Ferrovie e ANAS, ricapitalizzazione dell'ANAS), le amministrazioni centrali (con l'integrazione di numerosi capitoli di spesa rivelatisi incapienti, per lo più per obbligazioni assunte), gli impegni internazionali del nostro Paese (il fondo AIDS), la scuola e l'università, e molto altro ancora che non menziono per brevità. Le opposizioni hanno contestato e lamentato fino a poco tempo fa la natura elargitoria e disorganica delle nuove spese, l'abbandono della politica di risanamento finanziario, l'asserita scopertura del provvedimento. Le critiche sono ovviamente sempre legittime, ma a mio modo di vedere mai come in questo caso destituite di ogni serio fondamento. Il provvedimento, innanzi tutto, per le ragioni cui ho sopra accennato è tutt'altro che disorganico. Esso riguarda misure per spese obbligatorie, decisioni attuative di misure contenute nella finanziaria, provvedimenti concordati con le associazioni di categoria e con le parti sociali. Una manovra integrativa che si muove perfettamente in linea con gli indirizzi, i princìpi, le norme contenute nel DPEF 2006-2007 e negli strumenti di politica economica e finanziaria del Governo. E ciò vale anche per le argomentazioni che riguardano l'andamento della finanza pubblica. Ricordo che in tutti o quasi gli anni passati a metà anno venivano approntate manovre restrittive finalizzate a correggere i conti pubblici, che quasi sempre si rivelavano peggiori del preventivato.

degli indici di normalità, preciso che la volontà e la decisione del Governo per quanto riguarda gli studi di settore e gli indici di normalità economica è che valgono la presunzione semplice, la non automaticità degli accertamenti

tese a migliorare il nostro *welfare* e a fornire una prima concreta risposta ai sacrifici sostenuti finora dagli italiani. Si tratta di una manovra da 6,5 miliardi di euro a favore dell'economia e delle fasce deboli

interviene in favore dei Comuni in maniera significativa, ma ancora - a nostro avviso - non soddisfacente, stabilendo la possibilità per le Amministrazioni virtuose, cioè quelle che hanno

vero e proprio premio, riconosce il merito dei Comuni che hanno contribuito a conseguire gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica. E credo che anche in futuro il Parlamento e il Governo debbano procedere in questa direzione, incentivando il rispetto della legalità prima di tutto da parte delle istituzioni locali.

segnale che successivamente andrà sviluppato. Si tratta comunque di una prima parziale risposta alla grande domanda di sicurezza che viene dalla popolazione. Vi è inoltre lo sblocco del cuneo fiscale, esteso anche a banche e assicurazioni, senza aggravi sulla finanza pubblica, la rimodulazione dell'IVA sulle auto aziendali e i fondi alle imprese, che costituiscono un altro capitolo decisivo delle politiche di sviluppo. Ci sono gli studi di settore e, al riguardo, ringrazio il Sottosegretario per la precisazione che ha reso. Viene recepito in questo provvedimento molto opportunamente l'accordo tra il Governo e le categorie di rappresentanza delle imprese, accordo per la cui conclusione ha molto lavorato anche questo ramo del Parlamento, in particolare la maggioranza. Si è stabilito che gli indicatori di normalità economica, oltre che gli studi di settore, previsti per il periodo di imposta 2006 e fino alla loro revisione, abbiano natura sperimentale e valenza di prescrizione semplice fino al 2009. Dunque, finalmente è chiarito che l'onere della prova in caso di accertamenti è a carico dell'amministrazione finanziaria. Anche questa era una misura attesa che, sono convinta, agevolerà la ripresa del rapporto con quelle categorie economiche che si erano sentite penalizzate dalla legge finanziaria. La disponibilità al confronto la parte del Governo, sostenuta e chiesta da questa maggioranza, si è dunque tradotta in atti concreti.

nella discussione, il senatore Legnini, che se possiamo varare un provvedimento di spesa in questo momento, nella direzione che abbiamo detto, tutto ciò è possibile perché il governo Prodi ha avuto il merito di aver collocato il risanamento dei conti pubblici al primo posto della sua agenda politica, avendo ricevuto in eredità dal Governo precedente l'uscita dai parametri di stabilità fissati dall'Unione europea, un innalzamento della spesa pubblica e un rinvio dell'applicazione della riforma pensionistica al 2008. La dura polemica di oggi da parte del centro-destra sul superamento dello scalone avviene - a mio modesto parere - a scoppio ritardato. Se la riforma delle pensioni era una priorità, mi chiedo perché sia stata rinviata dal Governo Berlusconi.

possibile anche perché l'Italia è tornata a crescere dopo anni di stagnazione, uscendo dall'emergenza dei conti pubblici. Extragettito che, in quanto dovuto anche alla crescita della nostra economia, è merito del lavoro di tanti cittadini, imprese e istituzioni locali. Insomma, tutto il Paese ha il merito di questa ripresa della crescita, non soltanto il Governo per le misure rigorose assunte con coraggio nella finanziaria 2007. 2007. Il Governo in ogni caso intende rispettare gli impegni assunti con l'Europa nell'ambito della procedura di disavanzo eccessivo. Infatti, solo una parte dell'extragettito è impiegata per misure specifiche a sostegno delle classi più deboli e più precisamente quelle che sono le maggiori entrate strutturali. strutturali. L'accusa dell'opposizione di aver aumentato la pressione fiscale per sostenere una politica di spesa che peggiora i saldi di finanza pubblica è del tutto strumentale. la riduzione della pressione fiscale registrata nel periodo dal 2001 al 2006 (dal 41,3 per cento rispetto al PIL del 2001 al 40,6 per cento del 2005 secondo i dati ISTAT), obiettivo politico di assoluta rilevanza per l'Esecutivo di centro destra, come è stata finanziata? La riduzione delle imposte si può coprire solo con riduzioni di spesa, ovvero con gli effetti positivi di una maggiore crescita: se aumenta il PIL, aumentano le entrate, secondo un'elasticità che generalmente è pari o una riduzione delle entrate riduce la pressione fiscale). Cosa è accaduto tra il 2001 e il 2005? Il tasso di crescita reale del PIL si è ridotto. Quindi, senza crescita per effettuare una riduzione della pressione fiscale sostenibile, sarebbe stato necessario ridurre le spese. spese. Il saldo corrente è invece costantemente peggiorato, andando in negativo, e le spese sono costantemente aumentate: lo dimostra il *deficit* delle pubbliche amministrazioni sul PIL che dal 2,9 per cento del 2001 è salito al 4,4 per cento

imposte, ma anche i trasferimenti agli enti locali, i quali hanno dovuto aumentare i tributi di propria competenza per mantenere in equilibrio i propri bilanci, mantenendo così sostanzialmente inalterata la pressione fiscale complessiva. rispetto alle critiche dell'opposizione, possiamo affermare che la nostra è una politica economica alternativa ad una riduzione delle imposte in *deficit*: prima il risanamento, poi la riduzione del carico fiscale, anche perché la riduzione del carico fiscale, se fatta in *deficit*, non ha nemmeno effetti positivi sulla crescita. Gli operatori economici scontano infatti il fatto che prima o poi dovranno restituire ciò che viene reso loro al momento. Mi avvio alla conclusione, Il risanamento scelto da questo Governo e la riduzione del *deficit* del debito che ne consegue rappresentano una strategia di politica economica volta alla crescita e inoltre a fare fronte ad un ulteriore fenomeno negativo per i conti pubblici che non ha ancora sortito appieno i suoi effetti: la ripresa della crescita degli interessi sul debito. Quando si tratta di recuperare una fase di allarme economico-finanziario, il Paese segue le indicazioni della politica e ha dimostrato

è la capacità di raggiungere la meta finale del pareggio, secondo un percorso coerente di riqualificazione e di effettiva riduzione della spesa sin qui non completamente coerente e ben programmato. che gli strumenti che si stanno mettendo in atto portino in questa direzione, perché lo sforzo del 2006 non va vanificato per la mancanza di chiare scelte a sostegno dell'effettiva riduzione della spesa pubblica.

Presidente, quest'oggi l'Assemblea del Senato è chiamata ad esprimere un voto di fiducia al Governo utile a garantire la conversione in legge del decreto-legge n. 81 del 2007. Si tratta di un atto dalla forte valenza politica, di un provvedimento che è chiara manifestazione della volontà dell'Esecutivo di rispettare gli impegni assunti già all'epoca della campagna elettorale e che va in una duplice direzione (risanamento dei conti pubblici, politiche di sviluppo ed equità sociale) e che rappresenta una risposta alle aspettative dei cittadini, delusi per per gli ultimi corposi esborsi e in attesa che la morsa fiscale alla fine si allenti. Il decreto, infatti - lo ribadisco - ripartisce l'extragettito o tesoretto a chi ne ha maggiormente bisogno e a chi è da sempre oggetto particolare del nostro costante impegno, ovvero le categorie socialmente più deboli. In particolare, vorrei ricordare la previsione dell'aumento delle pensioni basse, con la destinazione di 900 milioni di euro per l'anno 2007, che andranno a beneficio di oltre 3 milioni di persone; cifra, tra l'altro, destinata a salire a 1.500 milioni nel 2008. In termini più concreti, ciò significa che ogni singolo pensionato riceverà tra 262 e 392 euro in più per il 2007, e tra 336 e 504 euro in più nel 2008, a seconda degli anni di contributi versati. Questa previsione rappresenta un primo passo verso quanto fortemente sostenuto, da tempo, da noi Popolari-Udeur sul tema fondamentale della riforma del sistema pensionistico. Tale progetto si sta perfezionando di concerto con tutte le parti sociali. Rispondono altresì alla medesima *ratio* le agevolazioni per il riscatto della laurea e la totalizzazione di contributi a favore dei giovani. Ancora, il decreto‑legge contiene importanti misure a sostegno delle imprese: lo sblocco della legge n. 488 del 1992, che accelera le procedure per l'erogazione degli importi ai programmi agevolati; i tagli al cuneo fiscale estesi a banche

qualche settimana fa. In quell'occasione ho avuto modo di sottolineare a gran voce la necessità di dare ascolto agli addetti ai lavori e alle associazioni di categoria per ricucire lo strappo che si era creato e pervenire a una soluzione immediata e condivisa. È dunque per me motivo di particolare soddisfazione l'inserimento nel decreto dell'intesa

alcuni dei punti qualificati della manovra, che contiene, tra l'altro, misure importanti di autorizzazione della spesa per il 2007: 80 milioni di euro per l'emergenza rifiuti nella vessata Regione Campania; 40 milioni per il servizio civile; 10 milioni per l'edilizia universitaria; 2 milioni per la lotta alle violenza sulle donne.

ne sia già a conoscenza, che il presidente Cossiga interloquisce direttamente con il Segretario generale del Senato nel decidere o meno se collocarsi in congedo, in missione o essere presente. Qualunque altra interpretazione, essendo ciò a conoscenza del Consiglio di Presidenza del Senato, serve a ricondurre i lavori che svolgiamo in quest'Aula verso

e il dottor Castiglia, è quella di interloquire direttamente con la Presidenza del Senato. Chiunque sostenga argomenti diversi, dichiara il falso. Venendo al merito della questione che ci interessa oggi, i senatori e le senatrici dell'Italia dei Valori non possono non dare il loro voto di fiducia su un provvedimento che arriva prima del tempo e siamo orgogliosi e contenti di poterlo affermare. Quando Quando si è insediata questa maggioranza, pensavamo che occorresse maggiore tempo per risanare i conti che il Governo e la maggioranza precedente ci avevano consegnato e quindi che un periodo, non dico di rigore, ma di attenzione ai conti pubblici e ai parametri europei, probabilmente

Paese: che saremmo stati rigorosi ed inflessibili sull'evasione fiscale. Probabilmente ciò ci ha messo in condizione di realizzare con minore necessità di tempo quello che avevamo preventivato: rimettere a posto i nostri conti, soprattutto in relazione all'ente sovraordinato nel quale abbiamo deciso di essere, cioè rispetto ai parametri europei, ed ottenere un gettito fiscale. Se parliamo di tesoretto o di extragettito è perché probabilmente

che in anticipo redistribuiamo ai nostri cittadini, a quella parte dei nostri cittadini che ne ha maggiormente bisogno, una parte di risorse, perché il risanamento è avvenuto. Questo è lo spirito con cui

(penso all'abbattimento dell'ICI e all'aumento delle pensioni minime) che stanno a significare per i cittadini della Repubblica italiana che l'attenzione ai conti ha dato i suoi frutti e che è cominciata la fase in cui qualche soldino (ma speriamo che siano sempre di più) può essere redistribuito, soprattutto verso quelle categorie che ne hanno maggiormente bisogno. Questo è il nostro concetto di solidarietà; è uno dei valori su cui si fonda questa coalizione, che potrà avere il difetto di discutere un po' troppo, ma che ha il pregio di saper decidere quando è il momento di decidere. E questo stiamo facendo oggi. In merito

rispetto alla larga maggioranza numerica, oltre che politica, della legislatura precedente; oggi al Senato lavoriamo, come è giusto che sia, con un po' di affanno.

e con la scadenza temporale, per la delicatezza e la rilevanza delle questioni ricordate prima, non vi era altra strada, per impedire che il provvedimento decadesse, che ricorrere al voto di fiducia. E noi siamo ben felici di dare la nostra fiducia al Governo su questo provvedimento.

a spendere ulteriori parole sulla devoluzione di questo cosiddetto tesoretto, alimentando in tal maniera il fiume di parole di cui sono stati investiti i *media* e i cittadini italiani da qualche mese a questa parte. Fiumi di parole che sono stati versati anche dagli esponenti di questo Governo, dal Presidente del Consiglio *in primis*, ma mai da questi ultimi ci è giunta una certezza. Quello che invece si è visto - e anche chiaramente - è la levata di un alto e consistente muro di gomma ove le legittime domande dell'opposizione, ma anche dei cittadini, sono rimbalzate. Più che a provvedimenti di alta finanza pubblica, sembra di assistere a vorticosi giochi di prestigio, in cui somme, dati, rilevazioni, stime, previsioni impazzano in un caos che annebbia e confonde. Siamo così giunti inevitabilmente e nuovamente all'atto conclusivo del dramma che ormai ogni giorno viene messo in scena da questo Governo; dramma che ci porta, insieme a quest'Aula tutta, ad essere sviliti, privati del nostro ruolo e della nostra funzione, svilendo e, quindi, privando del suo peso lo stesso popolo italiano che ci ha eletto. Il Governo, ponendo la questione di fiducia, l'ha giustificata parlando di necessità di proteggere l'equilibrio delle scelte operate attraverso questo provvedimento. Ma io allora chiedo: di quale equilibrio stiamo parlando? Questo maxiemendamento propone, come il testo originario, una serie disomogenea di provvedimenti in alcun modo legati a visioni di ampio respiro o a intenti riformatori. Mi chiedo, e mi rivolgo al Presidente del Consiglio: era così complesso permetterci di votare su questo provvedimento? Era così inconcepibile instaurare un legittimo e analitico dibattito sulla destinazione di denaro, frutto dei sacrifici imposti agli italiani? Ma partiamo della più semplice partiamo della più semplice delle domande e delle questioni: qual è l'origine precisa di questo fantomatico tesoretto? È effettivamente la tanto decantata manna dal cielo o solo frutto di un lavoro serio, duro e, diciamolo, anche alle volte impopolare, messo in campo dal precedente Governo? L'allora ministro Tremonti spesso fu accusato per la durezza dei suoi interventi in campo economico, interventi, quindi, alle volte impopolari, ma giusti e necessari, che di certo hanno nociuto sul momento all'immagine tanto del Ministro che del precedente Governo, ma i cui frutti possono essere oggi spesi per curare la profonda ferita che l'attuale maggioranza ha inflitto alla sua stessa popolarità attraverso un tasso di litigiosità che difficilmente si riesce a ricordare. A questo punto, infatti, è anche necessario essere sinceri, e se non riuscite ad esserlo voi, lo saremo noi al vostro posto dinanzi ai cittadini, a quest'Aula e a ciò che essa rappresenta. Non ammettete i meriti del Governo Berlusconi e allora dichiarate che ci troviamo davanti ad un palese errore nei vostri calcoli stessi in sede di finanziaria o anche che, in realtà, questo denaro non esiste, perché è solo frutto di una stima positiva in materia di entrate. Ma passiamo oltre, diciamo che vogliamo adottare il famoso proverbio: «A caval donato non si guarda in bocca», parliamo di cosa si vuole fare allora con questo denaro, che pure esiste, quindi. In linea di logica, un Governo di centro-sinistra, rispettando gli ideali di cui si è sempre vantato portatore, dovrebbe redistribuire queste somme alle classi meno abbienti, ai poveri, ai disagiati (e certo tra essi possiamo annoverare i pensionati titolari di pensioni al di sotto della soglia di sopravvivenza) e su questo non possiamo che essere pienamente d'accordo. Ma ci domandiamo, provvedimento alla mano, perché non sia stato utilizzato tutto il tesoretto come ammortizzatore sociale per operare una seria ed omogenea riforma del sistema pensionistico, come ci chiede l'Europa. La risposta è sin troppo semplice da dare: ciascuna delle molteplici e diversificate componenti politiche di questo Governo ha ben pensato di pagare ai propri "clienti" il prezzo richiesto. Vorrei ricordare che la reale equità sociale passa prima di tutto attraverso una reale riduzione del debito pubblico. Lo ricordo solo perché, di sicuro, è una certezza acquisita e condivisa. Anche alcuni storici dell'economia, alcuni grandi riferimenti europei hanno chiaramente spiegato che la priorità, in Italia, è ridurre è ridurre il debito pubblico per far si che si possa riguadagnare un'economia sana e dinamica. Aumentare le pensioni è una cosa bella, non definibile come priorità, ma noi, da sostenitori di uno Stato sociale efficiente e credibile, e sensibili alle sofferenze e alle difficoltà di un popolo sempre più anziano, possiamo sposare la decisione presa dalla maggioranza e ci siamo resi disponibili al dialogo sull'incremento delle pensioni minime, andando contro le giuste e correttissime indicazioni della Banca centrale europea che invitava questo Governo a non sprecare tale inaspettata ricchezza ma, al contrario, a destinarla al risanamento dei conti pubblici del nostro Paese. Non possiamo, purtuttavia, avallare in alcun modo l'attuale testo, che si perde in una miriade di provvedimenti tampone che finiscono per rendere infruttifero, anzi completamente vano, questo tesoro. Come al solito, chi realmente ci rimetterà per le azioni sconsiderate di questo Governo sono i giovani, che non vedranno mai la loro pensione duramente guadagnata e, paradossalmente, le classi più deboli, su cui ricadrà il peso del *deficit* pubblico che il prossimo anno schizzerà alle stelle poiché nulla è stato fatto per ridurlo. Il Governo sta firmando degli assegni in bianco, assegni privi di copertura, assegni che verranno scontati da tutti i cittadini a vantaggio di pochi. È il Governo dei "vorrei ma non posso", dell'annebbiamento delle coscienze e dei conti pubblici. È il Governo che propone scene populistiche e di facciata per ovviare alle grame figure del suo *Premier* e della sua maggioranza, ciascuno dei quali ben arroccato sulle proprie inconciliabili posizioni, dalle quali pretendono di governare questo Paese; e con quali risultati lo vediamo quotidianamente. Si è tanto pubblicizzato il giusto taglio dei privilegi ai parlamentari, azione dai dubbi effetti mediatici, ma ora è necessario soprattutto parlare dei problemi veri, quelli seri, quelli che portano le famiglie a non arrivare alla fine del mese, quelli che richiedono coesione, stabilità e ampio consenso, che voi di certo non avete. Quindi, noi convintamente voteremo contro questa fiducia, nella speranza che stavolta qualche anziano senatore abbia già anticipato le proprie vacanze.

Presidente, dichiaro il voto favorevole da parte del Gruppo Verdi-Comunisti Italiani alla richiesta di fiducia posta dal Governo. L'opposizione ha criticato aspramente la richiesta di fiducia. Tuttavia voglio ricordare che il provvedimento è necessario. Si tratta di garantire finanziamenti per alcune opere infrastrutturali, in particolare nel settore dei trasporti, per le Ferrovie dello Stato e la viabilità ANAS. Vi era e vi è il rischio molto concreto di chiudere alcuni cantieri. Quindi ritengo che il provvedimento, almeno sotto questo aspetto, non si può negare fosse necessario. Come ricordavo, l'opposizione ha svolto un'azione molto dura. Mi sono chiesto, Presidente, se il motivo di questa opposizione così intransigente fosse sul merito

del cosiddetto extragettito o l'ammontare dello stesso, perché ritengo che l'opposizione dovrebbe mettersi d'accordo con se stessa. Abbiamo sentito in Aula in questi giorni, ma anche nelle passate settimane, chi ha affermato che l'extragettito è molto più elevato rispetto a quello certificato e quindi ci sarebbe un falso in atto pubblico nel bilancio dello Stato, e chi, per contro, sempre dall'opposizione, ha affermato che l'extragettito non esiste e quindi questo provvedimento sarebbe non coperto. Immagino, Presidente, che l'opposizione sia dovuta alla questione della copertura, perché sarebbe difficile ritenere che l'opposizione così intransigente al provvedimento sia dovuta a questioni di merito. Come cercherò di spiegare dopo, infatti, vi sono questioni di merito molto rilevanti dal punto di vista sociale. che l'opposizione ha svolto un'azione riguardo alla copertura del provvedimento, portando anche dei rilievi legittimi sulla questione dell'assestamento e dell'articolo 1, comma 4, della finanziaria. Sull'assestamento, signor Presidente, alcune ragioni evidentemente ci sono. Tuttavia, non possiamo negare che l'extragettito è stato ampiamente documentato nel mese di novembre, a marzo con la relazione unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria e con le audizioni che il vice ministro Visco ha tenuto sia alla Camera che al Senato. Questo extragettito vale per il 2006 12 miliardi di euro, per il 2007 altri 12 miliardi di euro; anzi, ci sono già in più 2 miliardi di euro rispetto alle stesse previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria. La necessità di intervenire subito deriva anche dal fatto che il comma 507 della finanziaria non ha funzionato: i famosi tagli lineari non funzionano. Credo che questo Gruppo parlamentare, come ha fatto nella precedente legislatura l'allora Gruppo parlamentare dei Verdi,

da questa maggioranza. Sappiamo infatti, l'abbiamo visto ed è stato dimostrato, che il meccanismo dei tagli lineari non produce gli effetti sperati. Quindi, c'era il problema di rispondere ad alcune questioni lasciate in eredità anche dalla passata legislatura, per esempio la questione dell'IVA per le auto aziendali. Si dice poi che il comma 4 dell'articolo 1 legge finanziaria non poteva essere utilizzato a fini di copertura di questo provvedimento. Anche in questo caso vi sono certamente alcuni rilievi fondati, e a settembre vedremo quanto

finanziaria afferma che in quanto eccedenti e strutturali queste entrate possono essere utilizzate per ridurre il carico fiscale.

definiti incapienti, di soggetti che quindi non pagano le tasse; come si fa a ridurre le tasse a chi le tasse non le paga, perché ha redditi così bassi? Era l'unica operazione che poteva essere fatta. Credo pertanto che abbiamo agito bene, anche perché questo provvedimento ha una rilevanza sociale importante. Non si è d'accordo? Si dica Si dica che non si è d'accordo con gli interventi di carattere sociale contenuti in questo provvedimento: l'aumento delle pensioni minime, gli interventi sui giovani, il riscatto della laurea e la totalizzazione dei contributi. Si tratta pertanto di un provvedimento a sostegno dei redditi più bassi, per stimolare i consumi, un provvedimento che garantisce più sicurezza ai lavoratori giovani, ma anche che rifinanzia il "*bonus* bebé" (40 milioni

per le conseguenze drammatiche di quegli avvenimenti; non ricordiamo però che al G8 di Genova l'allora presidente Berlusconi aveva dichiarato che avrebbe aumentato gli stanziamenti italiani al fondo globale e che ciò non come dire, è un'eredita del passato Governo alla quale dobbiamo rispondere e dobbiamo far fronte. Infine, vi sono misure importanti per quanto riguarda le imprese, lo snellimento delle procedure per gli incentivi, l'abrogazione delle norme che prevedevano che gli incentivi dovevano essere considerati contributi in conto capitale e poi restituiti, la modifica delle norme sugli studi di settore e l'estensione del cuneo fiscale a banche e assicurazioni, i rimborsi IVA per le auto aziendali, come dicevo prima. Quindi, è un provvedimento giusto,

per la crescita del Paese e dell'economia, aprendo buone prospettive per la finanziaria: ridurre la pressione fiscale e sostenere lo sviluppo sostenibile e di qualità.

Signor Presidente, il Gruppo di Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo voterà a favore della fiducia al Governo sul decreto in discussione. Non è una fiducia data solo per lealtà all'Unione, ma esprime la soddisfazione del nostro Gruppo per i contenuti del provvedimento, che in gran parte condividiamo (come ha puntualmente specificato nel suo intervento il senatore Giovanni Battaglia), e anche per il metodo con il quale il Governo ha elaborato il decreto. La ripartizione del cosiddetto extragettito fiscale, infatti, pareva all'inizio che dovesse essere il risultato dell'accordo di una sorta di cabina di regia, quasi un "patto di sindacato" nel Consiglio dei ministri, abilitato a decidere per tutti. Per altro, questa cabina di regia, almeno fino a quando ha operato, non era stata neppure capace di quantificare l'entità effettiva delle maggiori entrate. I Gruppi parlamentari della sinistra hanno pazientemente ristabilito i princìpi di collegialità nella coalizione e le priorità nell'utilizzo del sovrappiù fiscale sono state il risultato di una decisione complessiva della maggioranza. A quella decisione complessiva i Gruppi della sinistra hanno partecipato presentando un'idea elaborata insieme, dopo incontri con le organizzazioni sindacali. La conseguente presa di posizione, nei confronti della Presidenza del Consiglio, di quattro Ministri espressione della sinistra nel Governo, ha consentito di quantificare con una relativa larghezza le risorse dell'extragettito e, soprattutto, di destinarlo anche alla ridistribuzione, così come non era chiaro nelle intenzioni iniziali. Si poteva fare meglio? Certo. Però la destinazione delle maggiori entrate, che derivano dal recupero dell'evasione fiscale, ha rispettato i vincoli dell'Unione Europea e, soprattutto, ha dato una prima risposta all'esigenza indifferibile di procedere ad una ridistribuzione del reddito, sia pure ancora limitata, a favore delle categorie sociali più svantaggiate e di migliorare la copertura dall'inflazione delle pensioni più basse. La ridistribuzione del reddito avviata con le misure in esame costituisce un'inversione di tendenza rispetto alle scelte insoddisfacenti della passata legge finanziaria. Certo, sarebbe stato meglio se alcune delle previsioni di spesa che hanno impegnato i circa 7 miliardi di euro del provvedimento finanziario fossero o escluse o limitate, per incrementare l'importo dell'aumento mensile delle pensioni più basse, quelle inferiori ai 650 euro, che il decreto fissa in 35 euro. È una misura ancora insufficiente, ma che comincia ad affrontare una gravissima emergenza sociale, che interessa più di 3 milioni di anziani alle soglie della povertà. Esprimiamo dunque un motivato consenso al provvedimento, che è una tangibile prova della ripresa economica in atto e dell'incisività della lotta all'evasione fiscale e costituisce una misura di ridistribuzione del reddito a favore delle condizioni sociali più svantaggiate. La finalizzazione delle risorse al *welfare* e ai redditi più bassi è stata dunque il risultato di un confronto non facile nella maggioranza, dove taluni sono troppo sedotti dai lamenti degli imprenditori e delle loro rappresentanze e particolarmente sensibili alle pretese della Banca centrale europea e del Fondo monetario internazionale. Queste posizioni hanno già influito negativamente sulla legge finanziaria dell'anno scorso, che doveva muoversi come ricordate - lungo le direttrici dell'equità, della solidarietà sociale e del risanamento della finanza pubblica e che non ha saputo tenere in equilibrio queste esigenze. Ne è seguita una forte delusione nei ceti popolari, come rivelano recenti indagini e sondaggi, e una delusione nel nostro elettorato di riferimento. I risultati delle elezioni amministrative, uniformi ed omogenei nella perdita di consenso delle forze del centro-sinistra, stanno lì a dimostrare che la causa di tutto questo è generale e non locale e dipende dalle misure messe in atto dal Governo con la passata finanziaria. L'Unione non può dividersi tra quelli che lavorano per portare voti e quelli che cercano il consenso delle autorità monetarie: entrambi questi obiettivi devono essere patrimonio di tutte le forze della coalizione. Serve quindi che le decisioni politiche fondamentali siano il prodotto di decisioni collegiali, maturate nell'insieme del Governo e condivise dall'Unione. Non ci sono pacchetti di controllo nella maggioranza che decidono le misure da adottare, e gli altri non devono fare altro che adeguarsi. Questa è la logica di un monocolore, non di un Governo di coalizione. Qui non c'è alcuna pretesa di dettare le scelte di Governo da parte della sinistra, ma semplicemente una richiesta di pari dignità nella coalizione. Noi ci batteremo perché il metodo del dialogo collegiale sia la regola aurea del Governo e dell'Unione. In questo provvedimento, pur con alcune difficoltà iniziali, la regola è stata rispettata e se ne vedono i risultati. Non si può dire la stessa cosa per le scelte in materia di previdenza, di lotta alla precarietà e sulla competitività, definite nel faticoso protocollo d'intesa col sindacato. Il Governo non era alle prese con un sindacato chiuso, corporativo e aggressivo, tutt'altro. Era evidente la comune intenzione di riformare la cosiddetta legge Maroni, quella sullo scalone, e la legge n. 30 del 2003, quella sulla precarizzazione del lavoro, in una direzione avanzata, innovativa e coerente con il programma dell'Unione, apprezzato esplicitamente dai sindacati su questi punti, al momento della sua elaborazione. Eppure sono passati mesi senza che si capisse qual era la piattaforma del Governo sulla previdenza e sul mercato del lavoro. In quella situazione, dove la collegialità del Governo sarebbe stata più incisiva, non c'è stato un confronto nella maggioranza, né condivisione degli obiettivi. Poi si è sostenuto che il Governo è ostaggio della sinistra, che questa non può tirare la corda, che servono alleanze "di nuovo conio", che ci vuole il *referendum* sulla legge elettorale per mettere la sinistra al suo posto. Il*referendum* è un'arma puntata sull'unità della coalizione. Non si può parlare di rafforzare l'unità del Governo tenendo la mano sull'elsa della spada del *referendum*. Si è sviluppata un'offensiva neocentrista, sostenuta da importanti organi d'informazione, che vuol fare della sinistra il capro espiatorio politico e sociale della crisi di consenso che attraversa il Governo. Noi siamo e resteremo leali col Governo e con la coalizione, non minacciamo nessuna crisi e semmai ci sentiamo minacciare la crisi. Votiamo i provvedimenti che condividiamo e cerchiamo di modificare quelli chi ci sembrano sbagliati e ci fanno perdere consensi e voti. Siamo convinti che i miglioramenti, rispetto al protocollo del 23 luglio scorso, sono possibili sulla previdenza, sono assolutamente necessari sul mercato del lavoro, dove le intese non alleggeriscono il peso del lavoro precario, e sull'incentivazione degli straordinari, quando esamineremo i provvedimenti di legge che li attueranno. Per noi il terreno è sgombro. Non ci sono veti o bandierine da piantare per motivi di ruolo o di visibilità, conta solo il merito e oggi il merito che vediamo sulla precarietà, sulla competitività, e anche su parti della previdenza non è convincente al punto da considerarlo il migliore degli accordi possibili. Se si vuole cominciare a limitare l'uso patologico dei contratti a termine non si possono consentire proroghe oltre i trentasei con la copertura di un sindacalista compiacente. La lettera della segreteria della CGIL al Presidente del Consiglio per la sottoscrizione del protocollo è per noi un importante punto di riferimento, ai fini dell'iniziativa parlamentare. Vedremo cosa dirà l'Italia dei pensionati, dei lavoratori dipendenti e soprattutto quella dei precari; aspettiamo l'esito della consultazione libera, democratica e vincolante, poi rifletteremo insieme. C'è però un problema politico che sarebbe sbagliato tacere e che può costituire l'occasione per mostrare la forza innovativa dell'unità politica della sinistra. Non possiamo chiedere cambiamenti delle scelte del Governo, come giustamente faremo alla ripresa, e poi vedercele ogni volta respingere nelle Aule parlamentari. Ogni volta si proporrebbe il dilemma: far passare tutto, o rompere. La sinistra, tutta insieme, deve allora chiedere un chiarimento politico al Governo, deve ricontrattare il programma che oggi viene disatteso e sbeffeggiato, come è avvenuto sui precari del tempo determinato. Non solo. C'è il problema della struttura e della composizione del Governo. Nuoce alla collegialità dell'Esecutivo e alla trasparenza della sua impostazione politica la composizione troppo numerosa, quasi pletorica del Governo: una sovrabbondanza di Ministri, Vice ministri e Sottosegretari (pochissimi dei quali della sinistra) che moltiplica le richieste, infarcisce le leggi di argomenti eterogenei, trasforma ogni provvedimento in un'affollata diligenza. Così non va. Il patto può e deve essere ridiscusso senza inutili drammatizzazioni per salvare l'alleanza di centro‑sinistra. Deve esserci pari dignità. Rifiutiamo il logoramento della sinistra e la falsa alternativa tra "rompere o accettare tutto" perché non c'è in questo Parlamento una maggioranza che possa escludere la sinistra. Allora, ridiscutiamo all'interno dell'Unione per avviare una seconda parte della legislatura più sobria e determinata, individuiamo un insieme delimitato di obiettivi impegnativi per tutti e una compagine ministeriale semplificata per realizzarli. Concluda, senatore mostra che questa è una proposta che nasce dal nostro impegno per l'unità della coalizione e per fortificare il suo consenso nel Paese.

dal senatore Ripamonti che chiedeva quali sono le motivazioni per cui la Casa delle Libertà voterà contro la fiducia su un provvedimento che incrementa

le motivazioni per cui parte di questa maggioranza voterà a favore della fiducia sul decreto al nostro esame. Le dichiarazioni che abbiamo appena ascoltato ci fanno davvero pensare e avere dei dubbi sul fatto che ci sia un'unità d'intenti sulla fiducia al Governo, visto che le dichiarazioni sono state assolutamente critiche per sia la composizione del Governo che le ultime iniziative in ordine all'accordo sulla previdenza, che, a quanto pare, dovrà essere consistentemente migliorato, a detta dei colleghi della sinistra.

pertanto che le sceneggiate che abbiamo visto in ordine a questo progetto di spesa avremo modo di rivederle.

reperite non certo con il recupero dell'evasione fiscale, bensì con l'aumento della pressione fiscale per incrementare la spesa pubblica. Quindi, il no a questa fiducia non è solo il no ad un decreto‑legge, ma ad una politica economica e fiscale di un Governo e di una maggioranza che si spacca in una schizofrenica politica fiscale in senso stretto,

discussione generale sul decreto, vorremmo parlare delle coperture o di altro, ma parlando in termini generali di fiducia o di non fiducia alla politica economica e fiscale di un Governo mi sovviene

diminuire la pressione fiscale in *deficit* o aumentare la spesa pubblica in *deficit*?

La politica economica di questo Governo, volta a porre in essere un determinato tipo di interventi, fa leva su una politica fiscale e di bilancio di spesa che incrementa sia la pressione fiscale, sia il *deficit* che la spesa pubblica. È una scelta. scelta. Rispondo ora a chi chiedeva: «Dite perché voterete no, oltre alle vostre contraddizioni interne». Voteremo no perché non siamo d'accordo con una politica di bilancio che vada ad incrementare la spesa pubblica:

che in termini di forti critiche nei confronti di un provvedimento che, invece di destinare buona parte delle maggiori entrate alla riduzione del debito,

il debito pubblico, la spesa pubblica e la pressione fiscale crescono: cos'è, questa, una forma di risanamento della finanza pubblica, di intervento costruttivo sugli investimenti per creare le condizioni perché in futuro ci sia una ripresa più consistente di quella che avete trovato, creata da altri, l'anno scorso, nell'esercizio 2006? 2006? Non possiamo assolutamente condividere il voto di fiducia su questo decreto, proprio perché rappresenta una

pur semplice logica di sistemazione delle questioni gravi e portanti che gravano sulla testa di ogni cittadino e di ogni impresa. Quindi,

Nord, non solo dà un voto contrario, ma si ribella fortemente allo spirito fraudolento - così lo definisco - nei confronti

Quindi, non possiamo che dare un significato rafforzato - non serve a niente, sappiamo che è un modo di dire - a questo no perché, da un lato, si incrementa la spesa pubblica, dall'altro si incrementa la pressione fiscale, che viene sostenuta in particolar modo dai cittadini del Nord, Nord, precipitando il Paese nel baratro di una non crescita, o perlomeno probabilmente di una crisi del settore produttivo privato, che c'è tutta ed è pronta a manifestarsi - pensiamo solo al settore degli immobili, ma potremmo riferirci a tanti altri tipi di attività

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo con esattezza che in questo momento l'ennesimo voto di fiducia sottolinea una difficoltà oggettiva non solo del Governo e della sua maggioranza, ma del sistema politico italiano.

ma l'uso che ne viene fatto - lo ricordava il collega Mannino - è strumentale e porta soltanto difficoltà al dibattito, che pure ci deve essere. Proprio a questo proposito, sappiamo con precisione che in questo momento non parliamo al Governo, non parliamo a questa maggioranza, ma parliamo al Paese, alla al Paese, alla situazione politica che dopo ottobre, dopo le questioni referendarie, si presenterà nel nostro contesto politico. Non possiamo però nemmeno sottrarci dal contribuire a restituire dignità al Senato della Repubblica e al Parlamento, signor Presidente, intervenendo in questo dibattito per rappresentare tutta la nostra acredine per l'ennesima forzatura politica che il Governo ci propone in questo contesto, senza permetterci di entrare nello specifico dei problemi per tentare di migliorare quello che questo bipolarismo sta distruggendo: un bipolarismo che nel nostro Paese Paese da bipolarismo politico è diventato bipolarismo elettorale e ora bilaterismo, dove tutte le forme di vita politiche, culturali, sociali, economiche, che sono al centro, vengono completamente distrutte e sottaciute. Gli interessi del ceto medio-basso, che diventa sempre più povero, i problemi delle nuove povertà che dovrebbero essere le priorità della nostre discussioni

non è solo di segno formale, signor Presidente, ma evidenzia una confusione all'interno dell'Esecutivo, tale da ingenerare anche ricadute di ordine istituzionale rispetto all'articolo 81 della Costituzione. La delicatezza della questione è stata riconosciuta da alcuni dei più sensibili e attenti componenti della stessa maggioranza, tra i quali il senatore Morando e il senatore Morgando. I "delitti finanziari" possono forse prolungare la vita di una maggioranza, ma minano alla base il fondamento di un'azione di Governo che appare sempre più orientata a soddisfare le esigenze preelettorali di una stagione politica ormai in corso di esaurimento.

Il provvedimento pone un problema di credibilità dell'azione di Governo di fronte ai cittadini. Un tesoretto che è mutato nella sua reale consistenza a seconda delle esigenze contingenti della maggioranza, a seconda dei Ministri, a seconda dei momenti e delle occasioni di propaganda. Non è in questo modo che potrà recuperarsi il consenso, ormai perso, del Paese e nel Paese, certamente più avveduto e smaliziato di fronte a un Governo che preferisce la logica delle promesse, delle illusioni, delle evasioni nelle ormai tante isolette di Prodi rispetto al principio di responsabilità di chi vuole concretamente affrontare i problemi delle persone, delle famiglie, dei giovani. Amici del Governo, non dobbiamo mai dimenticare che dietro ogni scelta politica dietro ogni scelta politica e del Governo, c'è una persona in carne e ossa. Questo dato di fatto si è ormai perso nelle valutazioni e nella sensibilità del Governo e di questa maggioranza. Il provvedimento sul cosiddetto tesoretto nasconde l'assoluta inadeguatezza dell'azione di Governo, che invece di fare seria autocritica rispetto al proprio operato, fortemente condizionato dall'area massimalista, si fa generoso dispensatore di consigli al prossimo, suggeritore finanche della Chiesa, dei vescovi, dei parroci, che dovrebbero, nelle loro omelie, a suo parere, correggere le storture e gli errori di tutti, tranne i propri. Siamo davvero alla farsa! Ci resta solo il conforto che il destino di questo Governo è ormai segnato. Non avete voluto ascoltare le ripetute sollecitazioni pervenute da parte delle istituzioni comunitarie e degli organismi internazionali (da ultimo, anche l'OCSE). Si segnalano, infatti, gli inviti affinché l'eventuale maggiore gettito nel 2007 sia per intero destinato alla riduzione del debito, contribuendo così all'accelerazione del risanamento rispetto al programma di stabilità. Avete, invece, pagato un dazio alla sinistra radicale

che ha messo in piedi l'ennesima opera di danneggiamento doloso del bilancio pubblico e del futuro delle giovani generazioni, quelle sulle quali verrebbe a gravare, in ultima istanza, il maggior debito che si creerebbe per effetto della rinuncia a destinare queste risorse alla riduzione della mole del debito pubblico. Sono convinto che di questo il Governo risponderà al Paese. Noi pensiamo ad

che il cittadino elettore possa scegliere oltre al partito e alla coalizione anche il candidato significherebbe restituire alla gente la rappresentanza popolare. Con questo sentimento, signor Presidente, esprimeremo un voto contrario alla fiducia ad un Governo che non rappresenta più nulla.

non chiede nuovi sacrifici agli italiani, ma distribuisce risorse: 6,5 miliardi di euro per interventi di spesa, a partire dall'aumento medio di circa 35 euro mensili per le pensioni basse. una misura che riguarda tre milioni e mezzo di pensionati. È una prima misura distributiva che, seppure insufficiente e parziale, comincia a dare un segnale e risposte ad una grave emergenza sociale che interessa milioni di anziani costretti al limite della povertà. In questo provvedimento, come hanno evidenziato i senatori Tecce, Bonadonna e Zuccherini, intervenuti nel dibattito generale (che, a nome del Gruppo, ringrazio per il lavoro svolto in Commissione ed in Aula), si interviene anche per garantire una migliore copertura previdenziale per i giovani lavoratori, così come vengono previste risorse aggiuntive per la scuola, l'università, il sistema del *welfare* e per le infrastrutture ferroviarie e stradali. Di rilievo è lo stanziamento per il Fondo mondiale di lotta all'AIDS, che porta finalmente l'Italia ad onorare un impegno internazionale. Il nostro Gruppo voterà la fiducia al Governo sul provvedimento in esame perché condividiamo le scelte di utilizzo delle maggiori entrate fiscali: 11,5 miliardi di euro, registrati già dall'anno in corso in virtù di un'efficace lotta all'evasione fiscale e di una più alta crescita economica; entrambi i fattori sono riconducibili all'azione e alle decisioni assunte dal Governo e dalla maggioranza. finanziaria - occorre ricordarlo - che non è stata certo indolore e che, anzi, ha chiesto agli italiani un indubbio sacrificio, volto a rimettere in sesto i malandati conti pubblici. Ancora una volta è toccato a noi dimostrare che cosa sia un'autentica visione complessiva del Paese e abbiamo prodotto una sterzata dopo anni di improvvisazione e di funamboliche politiche economiche e finanziarie. Le maggiori entrate fiscali, la gran parte delle quali di carattere permanente, non solo ci parlano di ulteriori riduzioni del debito pubblico, migliori di quelle previste in finanziaria, ma si proiettano sugli anni successivi e descrivono, anche all'estero, la realtà di un Paese che vuole scrollarsi di dosso l'immagine di ultimo della classe. Un allarmismo economico sulla tenuta dei conti è in questo momento del tutto ingiustificato e viene utilizzato dai grandi poteri economico-finanziari, nazionali ed internazionali, per impedire l'avvio di un vero progetto riformatore, così come previsto nel programma dell'Unione. Ed è proprio intorno a queste premesse che bisogna soffermarsi per capire dov'è che si inserisce la divaricazione tra gli obiettivi comuni e i nodi politici che invece ultimamente ostacolano un percorso che oggi potrebbe essere più agevole grazie alla situazione economica del Paese. Avevamo parlato, infatti, di fine della politica dei due tempi; avevamo parlato di crescita, equità sociale e rigore economico come di tre elementi che si tengono insieme e si giustificano l'uno con l'altro. Per noi quell'indirizzo era ed è giusto ed economicamente sostenibile, allora come oggi. Non sfugge a nessuno il legame coessenziale che tiene insieme il provvedimento che oggi poniamo ai voti con il DPEF e, in ultima analisi, con la strategia complessiva in termini di politica economica e sociale. Per noi, questa discussione ha immediate ricadute sulla vita quotidiana delle donne e degli uomini di questo Paese. Sebbene il provvedimento oggi in discussione sia largamente condivisibile, le recenti proposte sulle pensioni, sul mercato del lavoro e sulla riforma degli ammortizzatori sociali rischiano seriamente di parlare una lingua altra, ben diversa da quella che, con tutte le difficoltà del caso, il Governo e la maggioranza hanno parlato sino ad oggi. Esprimiamo forte preoccupazione per gli accordi che il Governo ha proposto alle parti sociali. La nostra critica va al merito dei provvedimenti. Non siamo mai stati interessati a difendere interessi corporativi e particolaristici; è una pratica che lasciamo volentieri a quanti, nell'opposizione come in alcuni settori della maggioranza, si ostinano a perorare le cause di pochi in luogo del bene comune e del futuro stesso del nostro Paese. Il dibattito sulle pensioni è costruito sulle finzioni scientifiche e statistiche, opportunamente veicolate da quanti hanno interesse alla costruzione di un sistema bipolare che tagli fuori ogni possibile voce critica. Non è vero che i conti dell'INPS siano al collasso, o che lo sarebbero di qui a qualche decennio. Non si dice - non lo dice la grande stampa - che solo in Italia i contributi dei lavoratori servono a pagare moltissime misure di assistenza sociale che invece dovrebbero essere a carico della fiscalità generale. Allo stesso modo, è indicativa la facilità con cui si è rovesciato il significato del conflitto generazionale del quale sarebbero responsabili i pensionati e i pensionandi che approfitterebbero di vecchi privilegi alle spalle dei giovani. A rigor di buon senso, è la permanenza obbligata al lavoro di schiere di anziani, spesso meno motivati, meno formati e meno produttivi, che restringe gli spazi per i giovani. Se nel DPEF si ribadisce giustamente il peso della precarietà anche nella scarsa contribuzione, in special modo per i giovani e le donne del Mezzogiorno, la proposta del Governo, fatta salva qualche misura condivisibile, si allontana in concreto da questa analisi, lasciando praticamente immutata la legge n. I rapporti di lavoro a termine, in affitto, a progetto, persino la mancata abolizione dello *staff leasing*, disegnano un quadro diverso da quello in cui buona parte di coloro che ci hanno sostenuto continuano a credere. È che dire del limite di 5.000 pensionamenti annui per lavori usuranti? O della ventilata ipotesi di innalzare l'età pensionistica delle donne, che da sola rende l'idea del grado di regressione culturale a cui si è scesi? Infine, se nel DPEF si fa riferimento alla necessità di aumentare la produttività del lavoro e migliorare la competitività del sistema Paese, gli accordi ignorano queste premesse e fanno leva su conti che tengono fermi gli attuali livelli di produttività. A dirla tutta, signor Presidente, la competitività continua ad essere vista solo in termini di tagli del costo del lavoro. Penso, ad esempio, alla decontribuzione degli straordinari, tutto a vantaggio di imprese che hanno già beneficiato di altre misure, come il taglio del cuneo fiscale, mentre continuano a non fare la propria parte su ricerca, innovazione, formazione. Ma il rovesciamento della realtà è un esercizio che ha molti e autorevoli praticanti, come coloro che oggi rinnegano il programma dell'Unione e accusano le forze di sinistra di ricattare il resto della coalizione, forze di sinistra che non vengono neppure consultate su provvedimenti fondamentali per la vita del Paese. Non si tratta di rivendicare una delegazione parlamentare più o meno nutrita, ma di ricordare che esiste un mondo, oltre i palazzi della politica, da cui il Governo e parte della maggioranza rischiano di separarsi. Le ipotesi sulle questioni sociali abbandonano un riferimento importante, consegnano cioè alla marginalità subalterna il mondo del lavoro, del precariato, del disagio sociale, la platea degli esclusi dal lavoro, coloro che sono privi di casa o magari sotto sfratto. Sappiamo bene che tutto questo è anche il risultato di un dibattito che si svolge in forze politiche diverse dalla nostra, e che, più opportunamente, dovrebbe tenere fuori tanto la sinistra quanto il Governo che, se non pone un argine, di questo passo rischia di esserne travolto. Sappiamo anche, signor Presidente, che qualche singolo protagonista è alla ricerca di quella visibilità che i nuovi scenari sembrano negargli. Intanto, però, rimangono fuori da ogni considerazione tanto l'analisi seria e realistica delle cose (come i problemi della gente comune), tanto la cause che portano alla progressiva perdita di consensi del Governo e dei partiti di maggioranza. Qualcuno potrà anche consolarsi con la balzana idea di escludere la sinistra o magari di metterle la mordacchia, e concluderne che per tale via si costruirà un sistema perfetto, bipolare, politicamente correttissimo. Ma sarebbe un'illusione effimera, destinata a scontrarsi con la durezza della realtà. Potrà non piacere a tutti l'idea, ma la sinistra è e rimane il legame che l'Unione e il Governo conservano con tutto un mondo di cui non si può fare a meno. È per questo che Rifondazione Comunista-Sinistra Europea non si accontenta. Non l'ha mai fatto, non ha mai rinunciato a mettersi in gioco, proprio per tutelare non gli interessi particolaristici, ma addirittura per «farsi carico dell'insieme», per usare l'espressione di qualche autorevole collega. Ed, infatti, ci permettiamo di rilevare, oggi, in quest'Aula, che il quadro tratteggiato dagli accordi su Stato sociale e pensioni pare del tutto privo di un'idea guida, di un modello di sviluppo, di un orizzonte di largo respiro; ripercorre un canovaccio abusato e ormai logoro; non incide sulle notevoli e montanti disuguaglianze sociali; né sembra concorrere a definire una strategia che affronti finalmente il tema del Mezzogiorno e di quel dualismo territoriale che rende un caso unico nell'Europa unita. Gli accordi che il Governo propone, con il metodo del «prendere o lasciare» che offende anche la sovranità parlamentare, producono una paradossale contraddizione con quanto di buono è contenuto nel provvedimento di quest'oggi e nel DPEF. Noi non ci accontentiamo e faremo la nostra parte per invertire una tendenza, senza estremismi verbali, senza velleitarismi di maniera. Occorre lavorare per superare il passaggio stretto. Per noi l'alternativa non è più tra l'etica della responsabilità e l'etica dei valori, come pure abbiamo letto in questi giorni su importanti quotidiani. Non ci accontentiamo di questa contrapposizione, ma cerchiamo di risolverla in modo che un'etica non inghiotta l'altra. È la difficile strada che abbiamo liberamente scelto di percorrere, ben sapendo che potesse infastidire i progetti di chi tende a semplificare il sistema. Noi riteniamo che l'obiettivo di un Governo con la presenza della sinistra non possa essere esclusivamente la gestione del presente o la propria salvezza, ma è miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, la riduzione delle ingiustizie sociali e il rilancio delle grandi riforme sul tema dei diritti civili. Oggi votiamo con grande senso di responsabilità e convinzione questo decreto-legge. La nostra fiducia di oggi al Governo è un investimento sul domani, convinti che in autunno, attraverso un processo di partecipazione e mobilitazione democratica, si possa avviare quel cambio di passo nelle politiche del Governo, necessario per riprendere quella connessione con il popolo dell'Unione. Non ci accontentiamo di gestire il presente, ma vogliamo trasformarlo per dare a tutte e a tutti un futuro migliore. *(Applausi *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio subito esprimere la mia più profonda gratitudine ai colleghi della maggioranza perché in questi giorni di dibattito mi hanno dato personalmente una lezione che non ero riuscito a capire nei quarant'anni precedenti, nonostante - le assicuro, signor Presidente - buone, forse ottime letture:

Qualcuno dei colleghi della maggioranza ha chiesto, giustamente, perché l'opposizione vota no. Io mi pongo un'altra domanda: come fa questa maggioranza a votare sì? Le parole appena pronunciate dal collega Sodano sono un palese, forte avviso di garanzia al Governo. Nonostante questo, debbo anche esprimere la mia solidarietà allo sforzo che i colleghi della maggioranza hanno dovuto compiere, grazie all'arroganza, all'ignoranza e all'imperizia del loro Governo. Sforzo che ha visto contrapposti i due fronti della maggioranza. una maggioranza spaccata palesemente su due fronti: da una parte, i riformisti che si sono ovviamente preoccupati, caro collega Ripamonti, delle modalità di copertura

la sinistra radicale, mi rivolgo sempre al collega Ripamonti, che è entrata nel merito del provvedimento. Entrambi sanno, al di fuori di ogni ipocrisia,

il merito del provvedimento, ovvero la sinistra alternativa, l'unico elemento che li accomuna, è la certezza interiore che entrambi i fronti mentono a se stessi, a quest'Aula e al Paese. *Sine pudore*, menzogna *sine pudore*, ovvero spudoratamente. Signor Presidente, questo dibattito ha infatti non solo sulla base degli interventi dell'opposizione ma soprattutto sulla base degli interventi della stessa maggioranza, due fatti chiari: che si è commesso un falso in bilancio a dicembre e che commetterete oggi, attraverso un voto di fiducia, un delitto finanziario. Non lo dico solo io, che lo sostengo da mesi, ma oggi lo hanno dimostrato vari interventi dei senatori della maggioranza. Ricordo, e lo potete verificare nel Resoconto stenografico,

infatti, collega Morgando, che se non aveste compiuto il falso in bilancio a novembre, oggi sareste in minore difficoltà e non dovreste arrampicarvi sugli specchi per giustificare questo attuale delitto finanziario. Il collega Morando, come presidente della Commissione bilancio, è stato ineccepibile e chiarissimo sia nel riportare le posizioni dell'opposizione, di fatto citando espressamente le nostre pregiudiziali punto per punto, sia nel riportare le difficoltà della maggioranza, riconoscendo che per l'anno 2007 il problema esiste. State decidendo un aumento di spesa senza aver ancora apportato l'assestamento Mancano i numeri delle entrate rispetto ai numeri della spesa che scriverete con il vostro voto di fiducia. Quindi, questo delitto finanziario

L'articolo 81 è chiarissimo e questo decreto è contro l'articolo 81, è contro la legge di bilancio, è contro le procedure di uno Stato di diritto che dà certezza al bilancio pubblico, è contro le indicazioni del Fondo monetario, dell'Unione Europea e della Banca d'Italia ed è contro il buonsenso. Non lo dico io.

questa maggioranza interpreta le cose in modo diverso dall'opposizione perché ritiene di poter dire che il bilancio di assestamento che verrà fatto a settembre

qui in Aula ha detto che è contro l'articolo 81, contro il comma 4 della legge finanziaria; usa l'articolo 77 della Costituzione contro l'articolo 81. Non a caso, il collega Boccia nel suo intervento - forse non lo avete notato - ha detto che tutte queste sono posizioni oggettivamente indifendibili, anche se politicamente comprensibili. E allora, più che assolti per il fatto che non sussiste, a me pare che con il voto di fiducia di oggi siate rei confessi. Non si può dire, collega Villone, che è successo tante volte anche nelle passate legislature, perché è una chiamata di correità; non si può dire che chi ha una anzianità di molte legislature meriterebbe allora l'ergastolo. Potrei rispondere che, essendo alla prima legislatura, mi disinteresso di questo aspetto perché un reato è reato. Se ponete la questione di fiducia per derubricare il reato di stupro nella nostra Repubblica, ebbene, mi sentirei di dire esattamente le stesse cose perché quello state compiendo è uno stupro finanziario, alla Costituzione ed alle regole della contabilità dello Stato.

L'attenuante non può essere che lo stato di confusione mentale, che forse a settembre diventerà seminfermità mentale. Chiudo con una battuta: qualcuno ha citato Einaudi e oggi il collega Sterpa risponde a questo qualcuno sulla citazione di Einaudi. Il compito della politica è aiutare i poveri, quelli che rimangono indietro; aiutarli sul serio, non prenderli in giro, ma aiutare i poveri non significa accusare il Governo di centro-destra di aver fatto i condoni e dimostrare, come Governo di centro-sinistra, usando un termine caro al presidente Cossiga, di dare una valenza politica al trattino. Questo è un Governo di "condoni", non ai poveri, non a chi ha bisogno, ma state donandovi voi per avere tre o quattro settimane di vacanza e rivedervi a settembre, a partire dal punto che ha lasciato alla fine non ultimo l'intervento del collega Sodano. Ecco, collega Ripamonti, perché il Gruppo di Alleanza Nazionale vota no.

il Gruppo di Forza Italia voterà convinto contro questa proposta che ci avete fatto, il cosiddetto tesoretto, perché lo riteniamo gravemente lesivo per il Paese e soprattutto per i cittadini italiani. Preliminarmente mi sia consentito, molto brevemente, di rammentare alcuni passi della storia recente e di evidenziare la situazione attuale della finanza pubblica.

cento del 2005, di innalzare le pensioni minime a 516 euro e di avviare più del 50 per cento del piano delle grandi opere, realizzando così il cosiddetto contratto con gli italiani. La XV legislatura si è invece aperta con le risultanze della cosiddetta *due diligence*, che abbiamo ritenuto una vergognosa operazione partita dalla campagna elettorale e il cui scopo era quello di evidenziare un buco nei conti dello Stato italiano. Tuttavia, a breve distanza il Governo ha avuto modo di verificare che la situazione non era quella a suo tempo rappresentata, ma ben diversa. Per tali motivi e per effetto della legge finanziaria 2007 si è in sintesi determinato un notevole incremento della pressione fiscale e creato il cosiddetto e famoso tesoretto. Al contrario, sono elementi di preoccupazione la dinamica della spesa pubblica, ulteriormente aumentata rispetto al 2006, e l'incremento del debito pubblico, che ha raggiunto il 106,8 per cento del PIL. Tali dati di natura congiunturale confermano dunque che la fase di riequilibrio della nostra finanza pubblica non si può ritenere certamente strutturale, vorrei ricordarlo anche all'ottimo senatore Morando, che stamattina ha ripetuto più volte che le entrate sono strutturali; non è vero, senatore Morando, e mi sorprendo che una persona seria come lei abbia potuto affermare queste cose. Si comprende pertanto che quello suggerito dall'Unione Europea, che ha chiesto all'Italia di utilizzare il tesoretto per una riduzione del debito pubblico, sarebbe stato l'unico utilizzo davvero equo e non suscettibile di critica. All'aumento All'aumento certo della pressione fiscale si accompagna, infatti, la mancata azione di contenimento della spesa corrente primaria (e questo Governo si identificherà con l'incremento della spesa corrente primaria). L'assurdità di un dibattito incentrato sul tesoretto (perché è stata una discussione assurda), che in realtà è solo un minore importo del*deficit* inizialmente stimato per il 2007, dovuto, come è evidente, a una sottostima del gettito 2007, emerge poi chiaramente dalle posizioni assunte, rispettivamente, dal governatore della Banca d'Italia Draghi e dalla Corte dei conti. Ricordo che, in occasione dell'audizione sul DPEF, il governatore Draghi ha testualmente affermato: «Non esiste un "tesoretto" da spendere, l'extragettito fiscale dovrebbe essere utilizzato per ridurre il disavanzo e il debito. Il rischio, se no, è quello di dover fare correzioni in futuro, quando il ciclo torna ad essere meno positivo». Queste poche parole del governatore Draghi possono sintetizzare quello che l'ortodossia in politica economica consiglia. Anche la Corte dei conti, durante la medesima audizione, ha evidenziato che la destinazione prioritaria alla riduzione del carico fiscale del maggiore gettito porta a ritenere che la manovra correttiva debba trovare spazio nel contenimento della spesa. Tale obiettivo appare molto problematico e, devo dire, è una vera vergogna del vostro Governo. Emerge, pertanto, un'opinione unanime, volta a sottolineare come si stia attuando una politica economica, nell'ambito del Patto di stabilità e crescita, totalmente incoerente con il ciclo economico. Come più volte raccomandato dalle istituzioni europee,

Più rozzamente - ma, se mi consentite, più efficacemente - è stato detto che si stanno avvelenando i pozzi. Vi sono, inoltre, ulteriori effetti perversi nella scelta di procedere, prima, ad una sottostima del gettito e, poi, allo sperpero in maggiori spese. non voglio parlare - come, giustamente, invece, ha fatto il collega Baldassarri - di falso di bilancio, ma le cifre sull'andamento delle entrate sono già state rese evidenti come un vero falso di bilancio. L'accumulo del tesoretto, infatti, ha determinato, in sede di formulazione del DPEF, un'evidente, maggiore resistenza dei Ministri al taglio della spesa corrente. Ne è la dimostrazione l'articolo 7 del decreto, laddove, al comma 1, dispone il disaccantonamento di una serie di spese che erano state appunto rese indisponibili dalla legge finanziaria, in vista di una loro successiva riduzione (nell'ambito, cioè, di quella che dovrebbe essere la logica della cosiddetta *spending* *review*). L'esperimento, con singolare dilettantismo, alla prova dei fatti è risultato, quindi, fallimentare. Riteniamo che questo sia un avvicinamento ad una prova elettorale, perché, altrimenti, non avreste potuto comportarvi in tale modo. Ma - fatto ancor più grave - la retorica del tesoretto ha scatenato gli appetiti di quanti si sono seduti al tavolo del confronto sulle pensioni,

Praticamente, gli unici esclusi da tale tavolo sono stati proprio i giovani: ne è la riprova il fatto che parte della copertura della revisione dello scalone verrà dall'aumento della contribuzione dei parasubordinati e, in caso di mancati risparmi derivanti dall'accorpamento degli enti di previdenza, anche dei lavoratori subordinati. Le forze sociali, con la sinistra massimalista, hanno avuto facile gioco, forti dell'esistenza di tale *surplus*, per sostenere la non necessità di innalzare l'età di pensionamento e la capacità della fiscalità generale di sostenere, anche in futuro, gli oneri di una mancata riforma del sistema pensionistico. Ironia della sorte, meno di un mese fa, Veltroni, futuro *leader* del Partito Democratico, dichiarava a Torino che la destra insegue gli interessi egoistici dell'oggi, mentre la sinistra

Come diceva un tale, un politico pensa alle prossime elezioni, che si deve sentire vicine, mentre uno statista, alla prossima generazione: questa non è non è una dichiarazione di Veltroni, ma di De Gasperi, un politico un po' meno giovane, ma decisamente più esperto e saggio, quanto a senso dello Stato. Nel merito tecnico della copertura del decreto-legge, va puntualizzato come la concreta possibilità di utilizzare a copertura di nuove spese mere previsioni di maggiori entrate rappresenti un grave *vulnus* alle leggi di contabilità, che richiede, invece, una variazione normativa *ad* *hoc*, a garanzia della solidità dei mezzi di copertura, tale da escludere che mezzi di copertura di nuove spese possano consistere in semplici previsioni di maggiori

mese. Giova rammentare che l'unico, vero aumento delle pensioni in Italia è stato realizzato dal Governo Berlusconi, che decise l'aumento generalizzato ad almeno 516 euro al mese (1 milione di allora). Si giunge anche ad aumentare gli stanziamenti per le missioni internazionali, dopo avere polemizzato con la sinistra massimalista, che è lì incollata alle proprie poltrone, con ingiusta criminalizzazione dei nostri militari all'estero, impegnati in missioni di pace. Molte di queste disposizioni suscitano poi preoccupazioni per i loro effetti sulla finanza pubblica. Si pensi all'articolo Si pensi all'articolo 2, dove, tramite l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione, si consente ai Comuni di aumentare la spesa. Si tratta di un intervento censurabile, in quanto spesso è lecito dubitare della solidità contabile degli avanzi di amministrazione dei Comuni. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi avvio a concludere. L'operazione complessiva, condotta con la sequenza di quattro atti (*due diligence*, sottostima delle entrate, decreti-legge Visco-Bersani e finanziaria 2007, con aumento della pressione fiscale ai massimi, e la cosiddetta operazione tesoretto) hanno reso evidente come la gestione della finanza pubblica

(questa sì sarebbe stata una dimostrazione di vera equità fiscale e intergenerazionale), più onesta (dopo la truffa contabile perpetrata dalla *due diligence*), più corretta (per non creare aspettative depressive di maggiore tassazione a breve) più leale, verso chi si troverà a governare dopo di voi, una riduzione progressiva e tempestiva della pressione fiscale, via via che le maggiori entrate si manifestavano, evitando che il tesoretto stesso si formasse.

è inevitabile che, nella discussione che ne consegue, il merito del provvedimento occupi sempre una posizione secondaria. Tutti partecipano più al dibattito politico generale e sviluppano considerazioni, analisi, proposte che allontanano molto dal merito del provvedimento la nostra attenzione. Credo però che questo sia un modo

che con questo provvedimento ricevono un sollievo, seppure non abbastanza importante come vorremmo, ma comunque ricevono attenzione.

sullo stato dell'economia del Paese, della sua finanza, dimenticando (o almeno molti se ne sono dimenticati) che questo Paese è stato governato per cinque anni, fino ad un anno fa, da una coalizione di centro‑destra e che, fino a due anni fa, la stragrande maggioranza delle Regioni era governata da coalizioni di centro-destra.

cercare di fare uno sforzo per affrontare con attenzione le questioni che sono poste davanti a noi,

stabilito che oltre le tre principali direttrici di azione (equità, risanamento e crescita) era necessario aggiungere qualcosa di più concreto e di più efficacemente

ciò che gli faceva comodo per sostenere la sua tesi. Ma di risanamento c'era bisogno, tant'è vero che abbiamo adottato provvedimenti all'interno di un programma che lo stesso centro-destra aveva negoziato con l'Unione di rientro; abbiamo adottato misure a favore della crescita che, come ho detto, stanno cominciando a produrre effetti concreti, tant'è vero che abbiamo invertito la tendenza passando da una crescita pari zero a quasi due punti percentuali.

Considero, infine, importante, ancorché non ancora affrontato da un punto di vista parlamentare, l'accordo raggiunto con le parti sociali

ciò che è accaduto nel corso di questo anno. Nel mese di luglio del 2006, mentre discutevamo il primo provvedimento economico importante del Governo, Governo, una parte dei cittadini protestava; era una parte minoritaria, per la verità, perché la gran parte condivideva quel provvedimento, soprattutto nella sua impostazione iniziale. I sondaggi di allora, infatti (a chi va a guardarseli), erano molto più favorevoli per il Governo. Oggi siamo a luglio ed agosto del 2007 il clima è indubbiamente diverso; c'è una difficoltà che noi avvertiamo nel rapporto con il Paese e d'altra parte le elezioni amministrative ne sono state un segno evidente. Siamo convinti che un Paese grande e importante come il nostro non possa vivere alla giornata: il suo Governo e il suo sistema politico devono poter operare in un arco di tempo che consenta di dispiegare e attuare la sua linea, il suo programma nelle sue parti più significative. Dopo un anno questa legge, con i suoi contenuti economici e sociali, è una tappa importante di questo processo che noi stiamo attuando. per così dire, un richiamo ciclistico, dopo le tappe della montagna che abbiamo fatto durante la finanziaria del 2007, cominciamo ad affrontare qualche tappa di pianura, con la quale noi pensiamo di dare una parte delle risposte che non siamo riusciti a dare finora. Ripeto, l'accordo con le parti sociali sulla previdenza e il *welfare* è un insieme di misure che riteniamo utili ed adeguate per cogliere i tre obiettivi che ci siamo proposti di equità, risanamento e crescita. Questo siamo convinti serva anche per fare giustizia di un giudizio sommario e troppo affrettato sull'azione di Governo che consideriamo del tutto sbagliato per il merito delle cose che finora sono state realizzate, ma ancor più sotto il profilo più strettamente politico. Mi rivolgo a quanti danno per liquidata troppo in fretta e con superficialità la forza politica e l'insediamento territoriale dell'Unione e delle forze che la compongono in questo Paese. Attenzione: noi forse abbiamo sbagliato nel 2006 a considerare già vinte facilmente le elezioni e in crisi irreversibile la Casa delle libertà; il dato elettorale in parte ci ha smentito, ma lo dico soprattutto a noi del centro-sinistra: attenzione a non fare l'errore di segno contrario, a considerare ormai liquidata la nostra forza perché commetteremmo lo stesso errore che abbiamo commesso alla vigilia delle elezioni politiche. Non ci sono all'ordine del giorno prossimo nuove e diverse maggioranze. Occorre uno sforzo ulteriore, al quale noi tutti dobbiamo essere richiamati, di coesione politica per serrare le fila e affrontare, fra tutte le componenti del centro-sinistra, gli appuntamenti che ci aspettano. Noi del Gruppo dell'Ulivo, che rappresentiamo in Parlamento il partito democratico che sta per nascere, portiamo il peso e la responsabilità più grande, e su questo, così come nel sostegno all'azione di Governo, non mancheremo di confermare il nostro sostegno e la nostra azione determinata.

non dicono nulla nei confronti degli evasori. Mi ero portato anche il testo del catechismo da dare al presidente Prodi, se avessimo avuto l'onore di vederlo, ma sono sicuro che esiste, perché così dagli atti risulta. Per il resto, credo che dovremmo cercare di tirar fuori meno parole ermetiche. Dico questo perché abbiamo fatto la campagna elettorale parlando del cuneo

10,25, un ordigno di straordinaria potenza distrusse un'ala intera della stazione di Bologna.

che, nelle ore immediatamente successive e il giorno dopo con le manifestazioni a Bologna, toccarono profondamente il nostro popolo e il nostro Paese. Ci sono state indagini, c'è stata l'azione della magistratura, ci sono state condanne; quindi, l'azione dello Stato c'è stata...

su questa vicenda un filo di incertezza, di opacità. Proprio nel ricordo delle vittime e del dolore delle loro famiglie, voglio qui riaffermare che per il Senato della Repubblica sempre, a partire da queste occasioni, la ricerca della verità, fino in fondo, resta la difesa e il cemento fondamentale della nostra democrazia.

sentimenti profondi, che durano ancora, di cordoglio ai familiari delle vittime toccate da quella così tremenda tragedia e sottolineo l'impegno del Senato della Repubblica, di tutti i senatori della Repubblica, a voler operare nell'azione legislativa, nella nostra testimonianza al Paese,

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza. Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto

L'articolo 62 del nostro Regolamento prevede che: «Un Senatore può mancare alle sedute dopo aver chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea».

quale mi ha riferito - come avrebbe poi comunicato al Segretario generale - che lui non aveva autorizzato nessuno a mettere in congedo se stesso, dopodiché si è fatto togliere dal congedo. Le altre richieste sono state comunicate, per conto del presidente Scalfaro, della senatrice Montalcini, del Pininfarina, da parte del Gruppo Misto. Io credo che la lettera del nostro Regolamento preveda che questa richiesta venga fatta dagli interessati e non attraverso la Presidenza del Gruppo;

Dopodiché, compare un altro foglietto per cui anche i colleghi Barbieri e Bordon risultano in congedo. Ma noi vediamo oggi qui presenti i colleghi Barbieri e Bordon, come anche la senatrice Montalcini e gli altri che si sono, casualmente dopo la mia segnalazione, per coincidenza,

che in passato, in assenza di verifica, il numero legale possa esserci stato sulla base di congedi che gli interessati non avevano mai chiesto. E queste sono regole! regole! Io accetto - ormai le polemiche sono passate - che un Governo viva, o non viva, sulla base del voto a favore dei senatori a vita, ma mi verrebbe da ridere se vivesse, o non vivesse, sulla base di chi vota no,

perché, attraverso i Gruppi, i senatori, tutti i senatori, che hanno stessi diritti e doveri, partecipano alla vita del Senato. poiché lei, anche per la carica che ricopre all'interno del Senato, eletto dai senatori, ha una posizione autorevole, se pone il problema io convocherò la Giunta per il Regolamento, anche a partire da questo momento, se vogliamo innovare a questa tradizione e prassi continua del Senato. Possiamo approfondire il problema, per tutti i senatori,

preciso. Quest'oggi abbiamo iniziato la seduta senza una verifica del numero legale. Se si fosse verificato il numero legale, sarebbe stato conteggiato anche il congedo dei colleghi Barbieri e Bordon, senza che vi fosse neppure la richiesta scritta da parte del Gruppo.

Rossi Fernando, Rossi Paolo, Rubinato,

Costa, Cursi, Curto,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, venerdì 27 luglio a Milano è morto Giovanni Pesce, comandante partigiano, medaglia d'oro al Valor militare. Il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, nel conferirgli questa importante onorificenza il 23 aprile 1947, così la motivò: «Valoroso combattente garibaldino, lottò strenuamente in Spagna per la causa della libertà e della democrazia riportando tre gravi ferite. Il movimento di ribellione alla tirannide nazifascista lo trovò ancora ardito e instancabile partigiano alla testa dei Gap al suo posto di lotta e di onore». Giovanni Pesce era nato il 28 febbraio 1918 a Visone, in provincia di Alessandria. Ancora bambino con la famiglia emigrò in Francia. A quattordici anni iniziò a fare il minatore, a soli diciassette anni decise di andare in Spagna a combattere in difesa della Repubblica e si arruolò nelle Brigate internazionali. Rientrò in Italia nel 1940. Venne arrestato per il suo antifascismo e, dopo un anno di reclusione, venne inviato al confino di Ventotene dove conobbe quelli che saranno i Padri della nostra Costituzione e della nostra democrazia: Terracini, Longo, Ravera, Pertini, Secchia, Di Vittorio, Rossi, Bauer e tanti altri. Nel settembre 1943 fu tra gli organizzatori dei Gap a Torino; nel maggio del 1944, braccato dai nazisti, fu costretto a trasferirsi a Milano, dove assunse, sino alla liberazione, il comando del terzo Gap. È proprio a Milano che conobbe la partigiana Nori Brambilla, che sarà la compagna di tutta la sua vita e a cui oggi vogliamo far sentire tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto. Dopo la guerra, Giovanni Pesce continua a lavorare con dedizione per la costruzione della democrazia attraverso diversi impegni politici, civili, istituzionali: è membro del Consiglio nazionale dell'ANPI fin dalla sua costituzione, presidente dell'Associazione dei combattenti volontari antifascisti di Spagna; dal 1953, per oltre dieci anni, è consigliere comunale a Milano. Non condivide lo scioglimento del Partito Comunista Italiano e aderisce fin dalla sua costituzione (nel 1991) al Partito della Rifondazione Comunista. Ha scritto numerosi libri nei quali ha raccontato la sua esperienza di volontario nelle Brigate internazionali in Spagna e di partigiano. L'impegno dei suoi ultimi anni è stato tutto teso a trasmettere alle giovani generazioni i valori e gli ideali per i quali ha lottato per una vita intera, in particolare: i valori della Resistenza, la strenua difesa della Costituzione, la lotta contro ogni forma di intolleranza e di razzismo, l'impegno per la pace e contro le guerre. Oggi, nel momento in cui Giovanni Pesce non è più tra noi, vogliamo non solo ricordarlo come Padre della Repubblica e costruttore della democrazia di questo Paese, ma anche impegnarci perché il suo insegnamento non vada disperso e il suo esempio di vita venga portato a conoscenza delle giovani generazioni.

apre una nuova finestra"). Comunico che il Governo ha preannunciato la possibile adozione di decreti-legge nei prossimi giorni e l'intenzione di presentarli in Senato.